Onorevoli colleghi, la Conferenza dei Capigruppo riunitasi questa mattina ha approvato modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 23 dicembre. La settimana corrente sarà dedicata alla discussione dei documenti di bilancio. In relazione al numero degli iscritti a parlare, entro questa sera dovrebbe concludersi la discussione generale. In ogni caso le votazioni degli emendamenti avranno inizio a partire dalla seduta antimeridiana di domani e si concluderanno - insieme al voto finale con la presenza del numero legale sul disegno di legge finanziaria entro la seduta pomeridiana di giovedì 11 dicembre, per la quale non è previsto l'orario di chiusura. La votazione della Nota di variazioni al bilancio, le dichiarazioni di voto finali e il voto finale sul disegno di legge di bilancio anche questo con la presenza del numero legale - avranno luogo nella seduta antimeridiana di venerdì 12. I Gruppi di maggioranza hanno ceduto proporzionalmente 45 minuti al Gruppo del Partito Democratico. In apertura della seduta antimeridiana di domani sarà commemorato il 60° anniversario della Dichiarazione dei diritti dell'uomo. Successivamente potranno intervenire i rappresentanti dei Gruppi per cinque minuti ciascuno. Come già preannunciato, all'inizio della seduta pomeridiana di domani la Presidenza ricorderà la figura del nostro collega scomparso, senatore Luigi Scotti. Per quanto riguarda i lavori della prossima settimana, l'Assemblea tornerà a riunirsi nel pomeriggio di martedì 16 dicembre per l'esame del decreto-legge in materia di disagio abitativo, approvato dalla Camera dei deputati. Sarà inoltre discusso - sempre la settimana prossima - il decreto-legge in materia di emergenza rifiuti in Campania, ove approvato e trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati. Su tale provvedimento i Gruppi di maggioranza hanno ceduto proporzionalmente 30 minuti al Gruppo del Partito Democratico. Mercoledì 17 dicembre, alle ore 17, si svolgerà al Quirinale la cerimonia per gli auguri natalizi al Capo dello Stato. Pertanto, la seduta pomeridiana avrà inizio alle ore 18,30. Nel corso della prossima settimana è previsto l'esame della mozione Rutelli sulla pirateria in Somalia e delle mozioni D'Alia e Giambrone sull'integrazione scolastica dei minori stranieri. Per i relativi dibattiti si è proceduto all'armonizzazione dei tempi. Il calendario della prossima settimana prevede inoltre l'esame del disegno di legge collegato recante delega sulla produttività del lavoro pubblico - per il quale si è proceduto alla ripartizione dei tempi, ai sensi dell'articolo 126-*bis* del Regolamento nonché del disegno di legge di ratifica del trattato di Prum sulla cooperazione transfrontaliera e il contrasto alla criminalità. I lavori dell'Assemblea proseguiranno nella settimana prima di Natale nella giornata di lunedì 22 dicembre, con seduta antimeridiana e pomeridiana,

nonché della relazione della Giunta delle elezioni sull'elezione contestata del senatore Nicola Di Girolamo e delle mozioni Cabras in materia di politica estera e Micheloni sugli italiani nel mondo.

all'assunzione di impegni, all'invito a trovare tavoli di dialogo, alla sollecitazione a far cadere steccati e barricate nell'interesse comune, dei cittadini. Sembra quasi un paradosso che poi l'atto concreto del Governo, con cui ci si preoccupa anche della giustizia, contempli esclusivamente dei tagli considerevoli proprio al comparto giustizia. È, quindi, un vano parlare parlare di riforme che si annunciano come *spot*, ma di cui non si conoscono i contenuti, di assoluta priorità per il Paese, di necessità dei cittadini di avere un servizio a livello degli altri Paesi europei: dobbiamo invece apprestarci a votare una legge di formazione del bilancio annuale che comporta una riduzione di spesa per la missione giustizia pari a 340 milioni di euro.

nell'arco di un triennio con un'estensione pari al 40,5 per cento delle risorse destinate alla giustizia. Noi, in particolare, troviamo nel documento che ci apprestiamo a votare 181 milioni in in meno per la missione giustizia; 81 milioni in meno per l'Amministrazione penitenziaria; in meno per l'organizzazione della giustizia civile e penale; 5 milioni in meno per la giustizia minorile e 43 milioni in meno per l'edilizia carceraria.

ben sapendo che non esistono riforme che possono essere fatte a costo zero. Eppure, noi sappiamo che i problemi che riguardano il settore giustizia sono indicati da tutti come prioritari. Ciò che sconcerta rispetto a questa situazione numerica così pesante e così impeditiva di qualunque progetto d'intervento normativo è è il dato che riguarda il personale. Sappiamo benissimo che le dotazioni di personale sono diminuite notevolmente, di circa un migliaio di unità ogni anno, e che attualmente vi è una scopertura di oltre l'8 Sembra un'anomalia, ma il dato della tabella 5 del provvedimento che stiamo per votare, illusoriamente indica un aumento del personale della giustizia: addirittura si parla di oltre 43.000 unità, esattamente 43.402, ossia più di quelle attuali. È soltanto un'effimera voce, in quanto non si è fatto altro che accorpare in un'unica voce anche gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari. Ripeto, si sono prese due voci,

con una progressione di depauperamento che ha fatto dire ai vertici

viene ad essere defalcato, in virtù delle norme che si sono susseguite, in virtù del divieto di *turnover*, oltre che dei tagli. Quindi, abbiamo una periferia

Ciò che lascia sconcertati è infatti come sia possibile che il personale amministrativo destinato al Gabinetto del Ministro passi da 207 unità al 31 dicembre 2008 a 283 unità al 31 dicembre del 2009 e che il personale destinato agli uffici ministeriali del dipartimento degli affari di giustizia passi da 268 a 330 unità. Assunzioni non se ne fanno, il *turnover* è bloccato, i tagli sono previsti, ma si aumentano le dotazioni degli uffici centrali del Ministero cento, togliendo personale agli uffici giudiziari distribuiti sul territorio. Questo è un fatto francamente sconcertante, avendo peraltro vissuto fino a maggio di quest'anno l'esperienza del Governo alla giustizia e sapendo perfettamente che si era alla copertura totale dei posti, ossia che non esisteva più margine per incrementare le dotazioni del personale agli uffici centrali. Ripeto, si era giunti alla copertura totale dei posti. Ora improvvisamente, da maggio di quest'anno, il nuovo Governo incrementa il numero del personale degli uffici centrali di circa il 30 per cento. È un dato così in controtendenza e così scandaloso che ci fa esprimere un giudizio totalmente negativo, per la parte che a me riguardava affrontare, sul provvedimento proposto dal Governo. *(Applausi

Signor Presidente, signori senatori e senatrici, avevamo a suo tempo avanzato il dubbio che la mancanza di un Ministro dedicato alla salute avrebbe consegnato la materia in mano al Ministro dell'economia e così è avvenuto. Di fatto, fino ad ora, le uniche iniziative degne di nota sono state i tagli orizzontali operati con la manovra di luglio e confermati con il disegno di che tolgono alla sanità in un triennio circa 9 miliardi di euro, per non parlare del taglio del fondo sociale e del fondo per le politiche familiari. La risposta alle nostre critiche è lo spauracchio del raddoppio nell'anno 2050 della spesa sanitaria; ma con la paura non si va da nessuna parte. Se la causa individuata è l'invecchiamento, quali sono i parametri esaminati? Un dato è certo: si diventa più vecchi, ma è cambiato il modo d'invecchiare, sono aumentati i livelli d'istruzione, viene praticata una maggiore prevenzione individuale, i livelli economici delle generazioni alle soglie della vecchiaia sono migliorati. Se non si vuole lasciare tutto all'iniziativa personale, il contenimento della spesa si fa mettendo in campo strategie per ridurre l'incidenza delle malattie croniche e degenerative, come tra l'altro ci chiede l'Europa. Perché negare, invece, che i tagli orizzontali, come quelli che sono stati fatti, colpiscono proprio i settori meno strutturati, come la prevenzione? A questo proposito, vorrei che ci venisse spiegato che fine faranno i piani di prevenzione impostati in questi anni e perché sono stati subito "avvicendati" il dirigente e il personale di maggiore esperienza, che bene avevano operato nella lotta al fumo, all'obesità, ai tumori, tanto per fare alcuni esempi. In un Paese come il nostro, dove le Regioni hanno costituzionalmente una grande autonomia in campo sanitario e dove si vuole attuare il federalismo fiscale, il primo atto di questo Governo è stato quello di mettere in soffitta il Patto per la salute. Con questo atto si chiedeva il rispetto del Patto di stabilità e il rientro da un deficit ormai decennale che rischiava di far affondare i bilanci di oltre sei Regioni; in cambio si dava certezza pluriennale nei trasferimenti delle risorse, per dare la possibilità di programmare investimenti e spesa corrente. L'aver fatto saltare tale Patto, l'aver tagliato i fondi all'Agenzia per i servizi sanitari, che avrebbe dovuto monitorare qualità e quantità della spesa, di fatto ripropone un sistema sanitario a diverse velocità, dove i diritti esigibili sono condizionati dal territorio in cui si vive. Con questi tagli, la ricerca, fiore all'occhiello dei Paesi avanzati, viene ulteriormente penalizzata: meno ricercatori giovani, meno fondi, meno qualità nel campo della cura e meno innovazione. Il taglio degli investimenti per l'edilizia sanitaria e per l'innovazione tecnologica degli ospedali e dei servizi viene giustificato con la decisione di facilitare l'utilizzo del sistema di *project financing*, senza un cenno alla complessità dello strumento e al fatto che alcune Regioni in Italia che l'hanno utilizzato non hanno avuto il risultato atteso. È mancato uno studio delle esperienze in Europa e uno studio degli strumenti legislativi atti a favorire il concorso del privato, senza determinare una privatizzazione spinta della sanità pubblica. Il taglio degli investimenti riduce innanzitutto la possibilità di riqualificare un sistema ospedaliero che per oltre il 70 per cento è vecchio e perciò inadeguato rispetto ai cambiamenti radicali operati nel sistema di cura in questo ultimo ventennio. Mancano gli investimenti nei servizi territoriali e questo mantiene più alta che in altri Paesi la spesa ospedaliera e costituisce un fattore un fattore di inappropriatezza della cura. Si vuole lasciare sulle spalle del medico di medicina generale, una figura su cui si fonda il nostro sistema sanitario, la responsabilità di fare rete per dare continuità di cura e appropriatezza alla cura stessa. Senza la rete, sarà difficile assistere in modo appropriato malati cronici, non autosufficienti, malati psichici e malati di tumore: tutte patologie che sono in aumento e a cui manca una strategia per rendere accessibili i servizi e il percorso di cura. Concludo, signor Presidente, sottolineando che è proprio la mancanza di strategie appropriate che fa aumentare la spesa. Il nuovo Presidente degli Stati Uniti ha detto nel suo programma che vuole dare la sanità a tutti, perché il benessere è ricchezza per una società.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, illustre Sottosegretario, il deterioramento recente del quadro congiunturale sta determinando in Italia, come in altri Paesi, un peggioramento spontaneo dei conti pubblici. Rispetto agli altri Paesi, però, l'Italia è in una posizione di indubbio svantaggio per il peso del suo debito di partenza e per il livello del deficit, anch'esso più elevato rispetto ad altri Paesi. A nessuno degli osservatori accorti sfugge che qualunque iniziativa che venisse percepita dai mercati come fattore potenziale di incremento del debito, si ripercuoterebbe ancor più sull'attuale differenziale tra i tassi italiani e quelli tedeschi, alla vigilia della scadenza di un importante *stock* di titoli di debito. Il fatto poi che la politica fiscale abbia in Italia minori margini di intervento costituisce un'ulteriore circostanza avversa nel corso della fase attuale. Abbiamo, infatti, una leva in meno per combattere la crisi rispetto ad altri Paesi, oltre che limitate risorse per fronteggiare il bisogno crescente delle fasce sociali più disagiate. Restiamo fiduciosi che, anche in virtù degli interventi di recente messi in piedi dal Governo per sostenere il sistema creditizio, le tensioni e gli allarmi che i risparmiatori e le imprese hanno percepito possano rientrare, salvaguardando il risparmio ed assicurando il credito necessario al sistema imprenditoriale italiano. Questo quadro di oggettiva criticità non rappresenta per la maggioranza un alibi per non mettere in essere politiche di bilancio espansive, né un alibi per negare livelli di sostegno al reddito delle famiglie in maggiore difficoltà. La scelta di non creare ulteriore debito parte dalla considerazione, finanche banale, che il rimedio alla recessione non può consistere nell'esporre il Paese - che ha il terzo debito pubblico del mondo, con un onere che supera ormai gli 80 miliardi di euro all'anno - al rischio della bancarotta. Per questo la strategia di questa manovra, che assume politiche di rigore del bilancio per riscuotere crescente credibilità ed affidabilità nei riguardi degli investitori, è la stessa dell'Europa: risanamento e sviluppo, come facce di una stessa medaglia. Di conseguenza, mentre la finanziaria smette di essere un veicolo *omnibus*, com'è stato in questi anni, ed assume correttamente il proprio contenuto tipico, altri strumenti legislativi si apprestano a farsi carico delle iniziative di sostegno dello sviluppo con necessarie azioni anticicliche. A tale riguardo, credo che sia degno di nota l'ultimo decreto, il n. 185, in esame alla Camera, che concentra importanti risorse su misure strategiche, di rapido impatto e naturalmente sostenibili dal punto di vista della finanza pubblica. al *bonus* per le famiglie: crediamo che l'immediatezza dell'impatto sui consumi di questa misura sia un fattore da apprezzare, al pari dell'alto contenuto sociale di questo intervento destinato alle fasce sociali l'intervento sui mutui per l'acquisto della prima casa, bloccati ad un tasso del 4 per cento; il blocco delle tariffe per le forniture abituali; la concessione di tariffe agevolate per le forniture di energia elettrica e di gas per le fasce sociali deboli. La stessa possibilità di concedere mutui di soccorso per sostenere la natalità è degna di considerazione, perché incrocia la vocazione fondamentale della famiglia, che è la natalità. Uguale attenzione è riservata all'altra gamba del sistema, rappresentata dall'impresa, a cui sono riconosciute riduzioni di imposta per tre punti su IRES ed IRAP; la proroga della detassazione dei salari di produttività; l'irrobustimento del finanziamento della cassa integrazione in deroga, con l'allargamento delle tutele ai soggetti finora esclusi dalla protezione degli ammortizzatori sociali. E, da ultimo, ricordo l'IVA, che verrà pagata al momento dell'effettiva riscossione, insieme all'annuncio degli studi di settore per rimodulare gli indicatori di reddito agli effetti della congiuntura. Tra le azioni di sviluppo si impone poi il grande tema del Mezzogiorno, da cui non vogliamo sfuggire. L'Europa ci sollecita, com'è avvenuto settimane fa a Reggio Calabria, a proseguire politiche di coesione per corrispondere alle dotazioni finanziarie imponenti, programmate per il prossimo sessennio, oltre 100 miliardi di euro, che dovrebbero permetterci di ottenere quei parametri di coesione e di convergenza da tempo attesi. Ci riferiamo all'urgenza di rendere possibile un maggiore e più efficace coordinamento tra i piani operativi delle Regioni del Sud, per progettare azioni e misure realmente funzionali al potenziamento del capitale umano, al rafforzamento dei sistemi produttivi locali ed al superamento dello svantaggio strutturale che ancora pesa negativamente sulle potenzialità di sviluppo di quest'area del Paese. Ha ragione il senatore Nicola Rossi quando sostiene che il problema è concentrare le risorse su obiettivi strategici, badando alla crescita e all'efficacia della spesa.

corre il rischio di nascondere la vera questione che, da meridionali, dobbiamo affrontare, come ci ha autorevolmente ricordato il Capo dello Stato. È sicuramente legittimo rivendicare le risorse necessarie per lo sviluppo, ma in pari luogo è necessario diventare esigenti sulla finalizzazione dei programmi e sui tempi della loro realizzazione. Siamo certi - e su questo abbiamo il dovere di mantenere una speciale vigilanza Il FAS ha rappresentato in questi anni una sorte di polmone finanziario modulato e ricostruito sulla base delle delle necessità di erogazione effettiva della spesa. Ciò è avvenuto con il Governo Prodi e sta avvenendo con questo Governo. Per il Sud c'è senza dubbio un problema di quantità necessaria di investimenti, una questione di qualità dei flussi di spesa, che non possono alimentare circuiti di spreco e di improduttività, per restare alla fisiologia. Nel Sud c'è' bisogno di una nuova temperie, che punti sull'innalzamento delle virtù morali di quelle comunità come premessa ineludibile di ogni progresso sociale ed economico. Per quel che ci riguarda, noi accettiamo questa sfida. *(Applausi

Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, di fronte alla manovra di bilancio l'opposizione del Partito Democratico si è distinta per aver percorso la via più dialogante e capace di mettere al centro il contenuto delle proposte per aggredire la crisi.

dai vincoli di stabilità e risanamento che ci legano all'Europa. Abbiamo anche manifestato apprezzamento per la scelta del Governo di anticipare a luglio la sessione di bilancio attraverso la predeterminazione dei saldi di finanza pubblica, una decisione che interveniva nel solco di una visione più ampia di riforma della stessa sessione di bilancio, una visione che ci appartiene, così come anche ci appartengono la difesa e la valorizzazione di ruolo e prerogative del Parlamento, della trasparenza dei provvedimenti (tema, questo, un po' oscuro per la verità, a fronte di tanta materia della legge finanziaria), del rigore e della disciplina della spesa.

in questo dibattito sulla manovra finanziaria, la discussione sulla politica economica in un frangente di crisi storica come quello attuale, perché qui ed ora si doveva fare tale discussione senza viceversa frammentarla e polverizzarla in una molteplicità di provvedimenti. L'altra faccia di questa decisione del Governo è che l'Italia fatica a reggere il confronto con le manovre di aggiustamento che interessano gli altri Paesi. Sul versante dell'economia reale, ovunque sono coordinati interventi significativi che fanno leva congiuntamente su investimenti pubblici, stimolo fiscale, sostegno alla domanda interna e alle fasce povere o impoverite dalla crisi. Sconcerta invece, nel caso del nostro Governo, l'assoluta incapacità di raccordare l'innovazione di percorso, introdotta con la finanziaria, con l'eccezionalità della crisi, una crisi certo globale ma con effetti tanto più gravi in un Paese come il nostro, che in questi anni ha visto crescere le sue fragilità strutturali e tutti i suoi divari principali con una sostanziale stabilità soltanto di un unico dato, quello della crescita zero. In questo contesto esistono due problemi, che la maggioranza ostinatamente elude: un problema di metodo e un problema di merito. Sul metodo. Da tutta Europa il messaggio è quello di cooperare e fare leva sulle risorse di collaborazione nei Paesi e tra i Paesi. Al contrario, per il nostro Governo il problema principale sembra essere quello non di fare "con" ma "senza" il contributo dell'opposizione. È singolare come le nostre proposte vengano puntualmente tutte respinte, senza una vera interlocuzione. A me sembra un comportamento irragionevole, che dovrebbe essere corretto. Penso che tutti possiamo condividere le parole del presidente Ciampi, che la settimana scorsa in una sua intervista ci invitava a ritrovare lo spirito del 1993, a riportare il Paese ad una collaborazione vera che sappia generare fiducia, che veda dunque un Governo capace di superare la tentazione di operare in solitudine. Per quanto riguarda il merito, quello del Governo non sembra essere un piano perché largamente insufficiente. Non è capace di parlare al Nord, al cuore produttivo del Paese, alle imprese, ai lavoratori che rischiano di perdere il posto di lavoro senza una prospettiva adeguata di ammortizzatori sociali. Non è capace di parlare al Mezzogiorno, che ha bisogno di investimenti, di occupazione, di legalità. E non è capace di rispondere a bisogni sociali vecchi e nuovi e soprattutto alla crescente povertà. Il ministro Tremonti, intervenuto alla trasmissione «Porta a Porta», a proposito della *social card*, con un tono giusto e apprezzabile, ha chiesto collaborazione e considerazione per quello che vuole essere solo l'inizio di una sperimentazione sociale. Benissimo la sperimentazione, benvenuta, ma a me piace citare un motto che propone la Caritas della Campania nella presentazione di un rapporto sconvolgente sulla povertà: «Non dare per carità ciò che è dovuto per giustizia, non dare per piacere ciò che è dovuto per diritto». Di fronte alle tante famiglie in difficoltà, di fronte alle tantissime situazioni di sofferenza e di disagio, per esempio quelle che ci racconta la Caritas, di fronte alle storie di tanti immigrati, ma anche di tanti italiani precari che diventano poveri per la perdita di lavoro, di fronte al fatto che dopo tanti anni e tante discussioni non siamo ancora riusciti a fare una riforma degli ammortizzatori sociali decente, di fronte alle minacce gravi di questa crisi, la risposta nazionale non può esaurirsi in una risposta emergenziale, ma soprattutto deve rimettere al centro i bisogni fondamentali delle persone come diritti di cittadinanza. E per fare questo è necessario porci in modo nuovo e diverso la questione delle risorse necessarie per le politiche sociali. Di questo, a mio avviso, dovremmo discutere. La risposta a questa crisi per l'oggi deve saper guardare anche al domani, e guardare al domani, come ci insegna l'America, significa riconoscere gli errori gravi, come la guerra all'Iraq - Bush l'ha fatto, in Italia non l'ha fatto ancora nessuno -, ma anche il fallimento del neoliberismo, con tutto il suo *côté* di esagerata opulenza e di miseria, di finanziarizzazione dell'economia e del debito, di degrado della democrazia e ridimensionamento del *welfare*. Ripartiamo dunque dal nostro *welfare* per cambiarlo, migliorarlo con un grande sforzo creativo pari a quello che originò il *New Deal*, ma con un cuore pulsante, un cuore europeo la senatrice Carloni.

per certi aspetti è falsata da una condizione generale di incertezza sulle previsioni reali della nostra spesa pubblica. Faccio solo un esempio:

la somma algebrica ci dice che calerà, secondo le previsioni del Governo, l'onere relativo al servizio del debito. Se la pensassimo così, se abbiamo cioè di fronte questa previsione,

che le prossime scadenze sulle emissioni dei nostri BOT saranno la cartina di tornasole, ma non per giudicare la tenuta del nostro sistema che riteniamo anche noi noi al riparo malgrado tutte le voci artatamente messe in giro. Indubbiamente farà una differenza capire se siamo capaci di ottenere dal mercato una fiducia maggiore o minore rispetto agli altri Stati che con noi su questo stesso mercato sono elemento di concorrenza.

ragioniamo su indirizzi generali ampiamente consolidati. Il Governo, come ha detto intelligentemente un commentatore non più tardi di qualche giorno fa, si atteggia in tal modo: adotta una linea

L'incertezza che si associa alla prudenza e al rigore di queste ore non mette il Paese fuori da un'ondata di accrescimento delle condizioni di dubbio, di fatica, di crisi.

non si procede

Invece, ancora una volta, ci troviamo di fronte ad un atto compiuto e dobbiamo discutere in base a qualche impressione, a qualche giudizio raccolto qua e là sulla stampa e che noi cerchiamo di ricomporre in un disegno unitario. un disegno unitario. Non può essere questo lo stile con il quale la discussione tra maggioranza e opposizione trova linfa vitale ed anche la cornice giusta per un dibattito degno di questo nome e soprattutto per soluzioni efficaci a contrastare la crisi.

Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, pur non facendo parte della Commissione bilancio ho partecipato attivamente alle sedute della stessa per sostituire un collega impegnato nelle elezioni abruzzesi e per perorare, purtroppo inutilmente, signor relatore, la causa dei terremotati del Molise e della Puglia, di cui parleremo successivamente. Devo lamentare, per la prima volta nella mia breve esperienza di parlamentare, l'inutilità assoluta del Parlamento di fronte a serie proposte di modifica della legge finanziaria da parte dei senatori di ogni Gruppo. Ci si è trovati di fronte ad un muro, spesso silenzioso, di rifiuto assoluto di discutere e accettare proposte valide, anche senza previsioni di spesa. Le stesse assenze dei Ministri competenti - ormai è diventata una norma, signor Presidente - e del Presidente del Consiglio delegittimano il Parlamento, che non può assolvere al proprio compito di legiferare, anche in presenza di noti condizionamenti politici e partitici al di fuori di queste Aule. È il caso di sottolineare, signor relatore, che tutta la rivoluzione sbandierata prima dell'estate sui contenuti e la qualità della finanziaria 2009 non siamo riusciti a vederla, a parte la giusta regola di impedire una legge *omnibus*, che abbiamo approvato anche noi. Del cambiamento annunciato non ce ne siamo accorti, se non subendo decine di decreti-legge blindati e spesso contenenti norme appartenenti a materie che fanno a cazzotti tra loro.

È questa la rivoluzione? Sommate tutti i commi aventi per oggetto la manovra finanziaria 2009 e vi accorgerete che non siamo tanto lontani dalle ultime finanziarie del centrosinistra, che contenevano oltre mille commi. Per la prima volta la legge finanziaria è stata ridotta, in conseguenza del decreto n. 112 del 2008, ad una semplice operazione di tagli, escludendo disposizioni finalizzate direttamente al sostegno dell'economia e ignorando la necessità di attaccare la grave crisi con giuste con giuste politiche di bilancio. È paradossale, ve lo ha ricordato egregiamente stamattina il senatore Nicola Rossi, che nella legge finanziaria annuale non vi sia la nuova politica economica. Si tratta solo di tagli di spesa, spesso indiscriminati, nei servizi sociali, nei settori della scuola, della ricerca, dell'università e perfino della sicurezza. Incomprensibili anche i tagli nella sanità sui fondi essenziali destinati all'edilizia sanitaria nell'agricoltura. Si tolgono 459 milioni di euro al settore agricolo, signor Sottosegretario, in crisi terribile terribile da qualche anno. Gli imprenditori agricoli - lo sa bene il ministro Zaia che sui mezzi d'informazione ha lanciato l'allarme - non possono più sopportare un taglio degli investimenti, che qualcuno ha addirittura quantificato nell'83 Questo settore avrebbe bisogno di innovazione, crescita, sostegni. Che dire dei produttori di grano - qualcuno li ignora - e della situazione terribile dei nostri agricoltori del Sud e del Nord,

Credo che occorra rimboccarsi le maniche per far sì che anche al Sud sia presente uno stabilimento per la lavorazione della bietola.

E che dire anche

questo spettacolo che dobbiamo dare domani davanti a Palazzo Chigi quando ve l'ho ricordato in Commissione, nel decreto precedente e tante e tante volte?

fermo restando che avete anche il dovere di controllare la ricostruzione: perché noi molisani siamo gente seria e non vogliamo incorrere in incidenti come quelli che si sono verificati in altre Regioni. Non compete a me, compete a voi. signor Presidente, onorevole Sottosegretario, se entro il mese non verrà data una risposta, anche negativa, ma motivata, credo che anche la delegazione parlamentare del Molise dovrà prendere qualche decisione. Abbiamo sempre detto che vogliamo collaborare rispetto a queste situazioni; credo che il terremoto non possa essere di destra o di sinistra e rifiutiamo venga strumentalizzato a fini politici. Certamente tra qualche giorno il presidente Berlusconi andrà a portare un decreto di finanziamento. Noi lo vogliamo da quest'Aula, da questo Parlamento, e vogliamo verificare a che punto è la ricostruzione, anche con Commissioni di indagine serie, per vedere come sono stati spesi quei soldi. Ecco perché anche noi dell'Italia dei Valori vi diciamo che di fronte a questa crisi ci si salva insieme. Questa arroganza del Governo non va nella strada La nostra disponibilità al confronto è totale anche se volete assolutamente metterci da parte. Noi, però, di fronte ai problemi della nostra comunità, del Paese, offriamo il nostro contributo, perché noi non siamo un incidente della storia. Qualcuno di noi ha culture diverse. Certo, non siamo radicati in culture politiche, così come lo sono tante forze presenti in quest'Aula, ma non possiamo essere considerati l'incidente della storia degli ultimi dieci anni.

che noi definiamo dittatura della maggioranza. Sì, siamo in una perfetta democrazia, ma la dittatura della maggioranza è il cancro della democrazia. Lo ripeto, la gravissima crisi economica che ci ha ricordato ieri lo stesso Papa

e un'attenzione seria da parte del Governo verso tutte le forze politiche, sindacali e imprenditoriali, evitando di operare subdolamente per dividere queste ultime, soprattutto con la manovra finanziaria. Il Paese, ve lo ripetiamo, si salva tutti insieme perché la crisi è estremamente grave.

Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi senatori, se le intenzioni non sono nutrite dai fatti, rimangono intenzioni, al più buone intenzioni. È quanto caratterizza la politica per le infrastrutture contenuta in questo disegno di legge finanziaria per Dalle cifre del provvedimento in discussione emerge una realtà assai diversa da quella preannunciata dal Governo che aveva più volte manifestato l'impegno a contribuire allo sviluppo del sistema infrastrutturale. I tagli pesanti delle risorse destinate alle infrastrutture smentiscono clamorosamente le promesse fatte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che aveva garantito stanziamenti per il rilancio della legge obiettivo con risorse pari a 14 miliardi di euro nel triennio 2009-2011 e a 4,9 miliardi per il solo 2009. Il disegno di legge finanziaria non contiene alcun finanziamento al riguardo, così come non vi è traccia di alcuno stanziamento aggiuntivo per il Fondo opere strategiche; anzi, rispetto al 2008, vi è una diminuzione del 15,6 per cento e nessuna previsione per gli anni 2010-2011. I tagli di spesa generalizzati colpiscono il settore più delicato dei trasporti ferroviari e marittimi, i residenti delle piccole isole e dei territori periferici e i pendolari, impedendo di intervenire con efficacia anche in materia di sicurezza stradale e sottraendo risorse finalizzate ai controlli stradali. La verità dei numeri è questa ed è riportata nero su bianco nelle tabelle del disegno di Si pensi alle Ferrovie dello Stato: in base alla legge finanziaria per il 2008 erano previsti 3.500 milioni di euro; ora saranno 2.362. di legge finanziaria per il 2009 vengono tagliati anche i 15 milioni di euro destinati alla sicurezza ferroviaria. In questo taglio del 30 per cento degli stanziamenti alle ferrovie non c'è un euro in previsione di spesa per il completamento del Corridoio 5 da Milano in direzione Est. Non abbiamo capito come il Governo intenda far fronte a questo impegno strategico per il Nord e per tutto il Paese. In questo quadro si annunciano sacrifici per il trasporto locale. Gli utenti sono alle prese proprio in questi giorni con i nuovi orari e si annunciano tagli e proteste. Preoccupa, inoltre, il ventilato aumento delle tariffe ferroviarie. Una forte sottolineatura merita la riduzione delle risorse destinate all'ANAS che, in base alla legge finanziaria per il 2008, poteva contare per il 2009 su 1.560 milioni; saranno 1.205. Si gettano così le basi per una ulteriore e pericolosa contrazione delle politiche per la manutenzione e la messa in sicurezza della rete stradale e autostradale. Le risorse destinate ad ANAS e non impiegate per garantire il controllo e la vigilanza sulle concessioni autostradali sono state poi riassorbite nella convenzione, gettando ulteriori ombre sull'effettiva volontà da parte di questo Governo di richiedere con determinazione alle concessionarie la realizzazione degli interventi previsti e di quelli non ancora effettuati. Inoltre, sono stati cancellati i finanziamenti triennali assegnati al Fondo per la promozione del trasporto pubblico locale e i finanziamenti destinati ai sistemi innovativi per il trasporto pubblico locale. Per quanto riguarda la sicurezza stradale, non si può non esprimere preoccupazione circa la riduzione a 35 milioni di euro dello stanziamento destinato all'attuazione, alla valutazione di efficacia e all'aggiornamento del piano per la sicurezza stradale che, nella legge finanziaria 2008, ammontava a 53 milioni di euro. In più, sono ridotti a meno della metà per il 2009 i 15 milioni di euro destinati all'informazione agli utenti in materia di sicurezza stradale. Signor rappresentante del Governo, le domando se la sicurezza sulle strade sia per questo Governo solo una casella del gioco delle emergenze che si susseguono una dopo l'altra: le stragi del sabato sera, poi le morti sul lavoro, poi le tragedie dell'immigrazione, poi la violenza sulle donne e ora la condizione delle edifici scolastici. È una casella del gioco delle emergenze o è piuttosto - come deve essere - una sfida da vincere e da vincere sul serio? Così definito, questo disegno di legge non sembra francamente rispondere alle esigenze primarie del nostro Paese e lascia disattesi tutti i grandi di progetti di sviluppo infrastrutturale. Di fronte al dato inaccettabile della sottrazione definitiva delle risorse originariamente destinate alle infrastrutture del Mezzogiorno e all'incognita sull'entità e la consistenza dei fondi FAS, il comparto infrastrutturale ha registrato una spropositata riduzione delle risorse per circa 1.900 milioni di euro. Per concludere, signor Sottosegretario, colleghi, come si concilia la scommessa sulle infrastrutture, per un Paese più competitivo e per affrontare la crisi economica in atto, con una drastica riduzione degli stanziamenti? Non è fantasia il ricorso all'aiuto dei privati per il finanziamento delle opere pubbliche

se le intenzioni non sono nutrite dai fatti rimangono intenzioni. Anche per quanto riguarda le infrastrutture, l'Italia ha bisogno di fatti che sono invece contraddetti da questa legge finanziaria.

ha comunicato che, occorrendo provvedere, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nonché del parere della Giunta per il Regolamento espresso nella seduta del 7 giugno 2006, all'attribuzione del seggio resosi vacante nella regione Lombardia, a seguito della morte del senatore Luigi Scotti, ha riscontrato, nella seduta odierna, che il candidato che segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo della lista alla quale apparteneva il predetto senatore è Maria Alessandra Gallone. Do atto alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di questa sua comunicazione e proclamo senatrice Maria Alessandra Gallone. Avverto che da oggi decorre, nei confronti del nuovo proclamato, il termine di venti giorni per la presentazione di eventuali reclami. **Ripresa della Signor Presidente, l'altro giorno, in una trasmissione in cui si parlava di fisica nucleare, ho sentito un fisico ben più importante nel campo della fisica di quanto modestamente possa essere io nel campo dell'economia, citare Epimenide con riferimento

seguente paradosso: la finanziaria non dice nulla, ma tutti noi parliamo della finanziaria. L'unico modo per scardinare il paradosso è quello di negare l'assunto principale. Infatti, il «Io sono cretese, tutti i cretesi sono bugiardi» si scardina con una negazione dell'assunto principale, dicendo cioè che chi parla è bugiardo a prescindere dall'essere o no cretese.

La riforma del 1978 che aveva indirizzato, con la legge di contabilità, le modalità di produzione in Parlamento dei documenti finanziari era la cosiddetta riforma Stammati, che seguiva l'innalzamento del debito pubblico dei primi anni Settanta. Nel contesto di una democrazia parlamentare, essa induceva il Parlamento a dotarsi di uno strumento per evitare che la finanziaria

di Achille che non può superare la tartaruga. Infatti, quando la situazione si evolve così velocemente, impostare una politica economica senza tenere conto di quanto succede nel mondo e negli altri Paesi equivarrebbe a far correre un Achille che non può superare mai la tartaruga.

tre variabili sono sempre le stesse: le risorse disponibili, quanto destinare allo sviluppo e all'offerta e quanto destinare alle misure espansive e alla domanda. Ora, le risorse disponibili sono poche perché voi sostenete di averci lasciato i saldi a posto ma non ci avete lasciato nessun soldo. Quindi, con pochi soldi è difficilissimo fare una politica che attinga a risorse che sono non disponibili ma indisponibili. Con risorse indisponibili, l'unica misura che si può fare oggi è quella di determinare una politica di instradamento. Come instradiamo la politica?

con cui si realizza la comunicazione non ci permette più di fare una politica economica chiusa ma di determinarci in un dibattito sulla politica economica costante, che ha visto (e che vede) il Governo non soltanto lavorare sui saldi ma essere un Esecutivo saldo forte. Un Governo saldo e forte può, a questo punto, portarsi all'esterno cercando, ancora una volta, di perimetrare il pericolo dei prossimi 12 mesi

come una Nazione che sta facendo di tutto per comprimere quel fortissimo debito pubblico che determina quel forte *spread* tra il rendimento dei nostri titoli di Stato e il rendimento dei titoli di Stato di altri Paesi. A questo punto, l'unica cosa che possiamo fare è essere

forti e responsabili tanto che i documenti economici prodotti da questo Parlamento e proposti da questo Governo ci danno la forte sensazione che la situazione sia affrontata con la giusta determinazione e che il futuro è molto più roseo di quanto ci si possa aspettare.

*(PD)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Sottosegretario, affrontiamo la discussione del disegno di legge finanziaria in una fase del tutto straordinaria con una crisi dell'economia reale che colpisce le famiglie, i pensionati, i lavoratori a reddito fisso, ma anche tante piccole e medie imprese. Nel momento in cui si impongono scelte di priorità il Governo attua una serie di tagli di spesa, colpendo alla cieca, senza preoccuparsi di ridurre veramente gli sprechi né di accompagnare questi tagli con progetti di vera riforma e razionalizzazione della spesa, della quale il Paese avrebbe pur bisogno, producendo così l'effetto non già di migliorarne la qualità, non di favorirne risparmi virtuosi, bensì di mettere in difficoltà anche i settori dove alcune spese non sono né sopprimibili, né rinunciabili senza adeguati processi di cambiamento e di innovazione. È il caso dell'agricoltura. Occupandoci di questa tematica siamo ancora alla ricerca della sua traccia fin dall'approvazione dello scorso Documento di programmazione economico-finanziaria, quando di agricoltura, pesca e agroalimentare non venivano preannunciati interventi né tantomeno previsti stanziamenti. Lo stesso è avvenuto praticamente nel decreto-legge n. all'interno del quale non solo non sono state previste specifiche misure per il settore, ma anzi le missioni di spesa del Ministero hanno subito ingenti tagli. Sono, quindi, i tagli la filosofia ispiratrice delle politiche agroalimentari di questo Governo che con la manovra di bilancio infligge un duro colpo al settore. di tagli che influiranno sulla produzione, sul reddito degli agricoltori, sull'occupazione, sulla competitività, sull'innovazione e sulla modernizzazione del settore e, quindi, del Paese. I tagli in agricoltura che ammontano per il 2009 a 459 milioni di euro (pari quasi al 26 per cento) metteranno in discussione il contributo del comparto alla ripresa economica. Mentre la spesa corrente viene ridotta del 10 per cento, quella in conto capitale subisce una contrazione del 40 i programmi più importanti finanziati dal Ministero che riguardano il sostegno allo sviluppo e la sostenibilità dei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e dei mezzi tecnici di produzione subiscono un drastico taglio di 423 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate per il 2008. Di questi, 354 milioni ineriscono la spesa in conto capitale e, cioè, gli investimenti fissi, gli acquisti di terreni, i contributi agli investimenti delle imprese e delle famiglie. Riconosciamo, tuttavia, che il Governo non si è dimenticato di alcune misure, condivise e concordate, quali la stabilizzazione dell'IRAP agevolata ed altre proroghe per agevolazioni fiscali; ma non possiamo non sottolineare come questi provvedimenti, seppur importanti, siano insufficienti. Il rafforzamento del sistema agroalimentare ha portata strategica per lo sviluppo equilibrato di un paese come l'Italia, soprattutto adesso. Questo settore, che merita e che avrebbe bisogno di maggiore attenzione, registra purtroppo l'assenza di una strategia politica sui comparti dell'agroalimentare e della pesca. Non abbiamo visto, e non vediamo neanche oggi, interventi per lo sviluppo né per un loro reale sostegno. I provvedimenti che mancano, e che sono stati richiamati all'unanimità dalla Commissione agricoltura, dimostrano che anche nelle forze di maggioranza c'è la consapevolezza dell'insufficienza delle politiche messe in campo. Richiamo in particolare il Fondo di solidarietà nazionale che non è stato rifinanziato, vanificando una misura che viene considerata una delle più avanzate in ambito europeo e un formidabile aiuto al settore in un momento di particolare fragilità, accentuata dall'esposizione ai mutamenti climatici. per una migliore e più efficiente gestione delle risorse idriche, si taglino le risorse destinate al piano irriguo, oppure le risorse per sostenere il settore delle previdenze sociali per le zone agricole nelle aree sottosviluppate. Insomma, non vediamo politiche strategiche quando vengono elusi i temi del ricambio generazionale e dello sviluppo delle imprese giovanili e femminili. femminili. Non riscontriamo poi alcuna attenzione ai distretti rurali ed agroalimentari, che promuovono il territorio con la qualità dei prodotti e si ergono a difesa nelle emergenze.

presidente, adesso anche per la legge finanziaria possiamo usare la In estate la prima finanziaria, adesso la seconda, ma entrambe si dimostrano incapaci di dare una risposta seria e profonda alla crisi internazionale e, in particolare, alla specificità della nostra crisi strutturale, che espongono il sistema Italia a delle gravi conseguenze. Tutti i paesi avanzati hanno già avviato risposte forti, con consistenti e aggiuntive risorse pubbliche per sostenere la domanda, le imprese, le opere infrastrutturali, i redditi medio-bassi, le sacche di povertà e il sistema bancario. A luglio pensavate di fare un colpo di genio con misure veloci, a partire dal DPEF, impedendo oggi una finanziaria con norme sullo sviluppo. colpo di genio che ha prodotto un topolino in termini di sostegno alla crescita e un disastro con tagli rovinosi verso il ceto medio, la scuola, le imprese, l'agricoltura, il Mezzogiorno, la giustizia e la sicurezza. Adesso vi siete legati le mani con una finanziaria che sembra fatta a prescindere da quanto di drammatico nel frattempo è avvenuto nel mondo. Sembra la finanziaria de «La Bella addormentata nel bosco», tanto che siete stati costretti a ricorrere ad un decreto ulteriore (il n. 185 del 29 novembre scorso, che esamineremo), che utilizza di fatto poche risorse, le distribuisce in modo scriteriato, senza effetti sulla domanda e sulla crescita né alcuna ricaduta positiva sulle insopportabili ingiustizie sociali, di reddito e di territorio, presenti nel nostro Paese. Dovevate avere più coraggio per fare scelte diverse e mettervi in relazione con le risposte che il Paese si attende e che nel mondo si diffondono. In Italia niente di corposo. Certo, abbiamo il debito pubblico, ma avevamo anche un vantaggio, ossia quello di non dover sostenere le banche, perché non esposte come le altre nel circuito malato della finanza mondiale. Alle banche semmai dovevate chiedere un atteggiamento più serio, non chiedere rientri impossibili, come stanno facendo, nei confronti delle piccole e medie imprese, sottoponendole a gravissimi rischi senza che il contesto finanziario richiedesse un atteggiamento di questo tipo. niente di positivo e, come nel 2001, di fronte a questa ben più grave e strutturale crisi, lasciate il Paese solo a sbrigarsela con le sue difficoltà di fondo. Mi sembrate rassegnati a volare bassi e ad accettare livelli di PIL inferiori, anche nella caduta, alla media europea. Democratico abbiamo proposto un'altra strada, realizzabile, con un impatto positivo sull'economia e sulla società; abbiamo proposto di giocare sul rapporto deficit-PIL per liberare quest'anno un margine virtuoso di sforamento, compensato da un rientro definito attualmente, per fare cose altrettanto serie: sostenere il reddito medio-basso, le imprese e il Mezzogiorno. Mi soffermo sul Mezzogiorno: non avevamo occasione migliore di questa crisi per trasformare il Mezzogiorno da problema atavico, ormai strumentalizzato e retorico, in risorsa vera, dinamica, in affermazione, in rapporto inedito tra la dimensione della legalità e quella dello sviluppo. Sì, è il Mezzogiorno il luogo dove far ripartire la crescita complessiva del Paese; nel Mezzogiorno ci sono i più ampi margini di crescita, ci sono le risorse umane disponibili, ci sono degli effetti mediati che potremmo constatare in tempi velocissimi su tutta l'economia.

ma avete burocratizzato il meccanismo, facendo rientrare dalla finestra quello che noi del centrosinistra avevamo

fondi FAS non avete sfidato il Mezzogiorno o l'opposizione nel chiedere un utilizzo mirato, veloce, qualificato e produttivo nei confronti dei territori, delle aree e delle Regioni ma avete fatto una cosa un po' vigliacca: avete tagliato quei fondi. Sono stati tagliati per finanziare spesa corrente, spesa clientelare, spesa improduttiva; fondi che avete tagliato per destinarli non alle aree dell'Obiettivo 1, non al Mezzogiorno nella quota dell'85 per cento, ma ad altre aree territoriali, per altri obiettivi spesso non molto nobili e spesso inqualificabili. Abbiamo Abbiamo più volte sollevato tale questione, più volte vi abbiamo incalzato e continueremo a farlo anche con la presentazione di alcuni emendamenti in Aula. Vi chiederemo, in modo particolare,

che hanno bisogno di un differenziale virtuoso a proprio vantaggio per dislocarsi nelle aree sottoutilizzate. Vedremo se ci sarà una vostra disponibilità al confronto. In Commissione bilancio non avete dato alcun segnale positivo; eppure erano emendamenti per i quali vi era copertura; eppure sono emendamenti che potrebbero determinare un beneficio immediato e notevole. Ma la cosa ancora più beffarda l'avete fatta nei confronti della Sicilia: e non bastano la retorica e i sofismi che abbiamo ascoltato in quest'Aula da parte di un numero elevatissimo di senatori meridionali, in particolare siciliani,

E così, dall'inizio della legislatura, in attesa di una legge risolutiva, si sono sprecate le affermazioni di soddisfazione che sanno appunto di ambiguità, di retorica e nascondono bugie sui tagli certi che nel frattempo sono stati fatti. Avete giocato anche con il ponte sullo Stretto. Il Governo di centrosinistra aveva indicato un'altra priorità

voi avete cancellato queste risorse per coprire una legge i cui benefici (l'ICI e gli straordinari) andranno sicuramente nelle aree del Centro-Nord.

non ci fidiamo, ecco perché il Paese comincia a non fidarsi più di voi; ecco perché anche questa finanziaria è un'occasione mancata, un danno certo per il Paese e per il Mezzogiorno. Abbiamo fatto bene a presentare una relazione di minoranza, con proposte serie e fattibili che faremo valere in Aula e soprattutto nel Paese.

signor rappresentante Governo, colleghi senatori, voglio svolgere in questi pochi minuti una considerazione di carattere generale e due considerazioni di merito. Quella di carattere generale è ampia. Non sta certo a me ricordare a voi, e tanto meno al sottosegretario Vegas, come erano le leggi finanziarie fino a poco tempo fa, fino all'anno scorso:

di inquadrare la risposta pubblica che viene data attraverso le leggi dello Stato (in particolare con la legge finanziaria, ma anche con gli altri interventi realizzati), in maniera coordinata, ordinata

parti più consistenti con il decreto-legge n. 112 del 2008, addirittura prima della grave crisi finanziaria che si è manifestata nei mesi successivi, dimostrato lungimiranza e capacità di interpretare i fatti e gli eventi dell'economia in maniera assolutamente corretta e tempestiva.

che sembravano governare solo gli interessi delle Camere e non tanto quelli del Paese. Vi è stato quindi il tentativo di governare su un periodo di tempo effettivamente triennale, come il decreto-legge n. 112 cerca di fare, e non in modo fittizio tramite un bilancio di

uno degli elementi - parlo di metodo, più che di merito - che danno la certezza di una guida solida verso l'obiettivo che si vuole perseguire,

per le quali dobbiamo riuscire a intervenire in maniera concreta. Credo che il Governo l'abbia fatto in maniera assolutamente meritevole del nostro plauso.

per la quale in parte sono state accolte anche le istanze degli enti locali. La Lega, in particolar modo, aveva anche proposto di fare un passo in più, ossia di distinguere in maniera assolutamente netta da quelli non virtuosi, ossia quelli in grado di gestire le proprie risorse in maniera produttiva e capaci di controllare la propria finanza interna da quelli che invece non lo sono.

e credo che essi rappresentino un'importante novità rispetto al passato sia nel metodo che nei contenuti. Da molti anni in Parlamento discutiamo sui possibili rimedi ad una situazione che progressivamente si fa sempre più grave, fino a diventare insostenibile; mi riferisco al sovraccarico di decisioni e conseguentemente di stress e di tensione che la sessione di bilancio ha sempre comportato. Oggi il Governo ha deciso di presentare una finanziaria, che qualcuno ha definito *light*, leggera, ma che in questo difficile momento di crisi globale internazionale è l'unica finanziaria possibile. Una finanziaria che è stata votata alla Camera con un voto chiaro e senza ricorso alla fiducia. Per l'Italia è fondamentale oggi evitare di avviarsi verso quattro anni di crescita zero, consapevoli del fatto che per i due terzi la politica economica italiana dipende dalla BCE e da Maastricht. Allora sottolineiamo la portata innovativa di questo disegno di legge che si presenta molto ridotto rispetto al passato, che si sviluppa in tre articoli sostanziali: fissa gli obiettivi dei saldi di bilancio; dispone la proroga di norme di carattere tributario recanti regimi agevolati e incidenti sulla misura di aliquote o comunque sulla determinazione di parametri da cui deriva il *quantum* della prestazione; definisce l'importo delle risorse destinate ai rinnovi contrattuali e alle modifiche del trattamento economico del pubblico impiego, nonché l'importo dei trasferimenti destinati agli enti previdenziali. previdenziali. Dobbiamo fare una riflessione; tra i tanti problemi sociali ed economici, che la crisi finanziaria internazionale ha determinato, ce ne è uno che riguarda in modo particolare il legislatore, cioè il Parlamento, in Italia e in qualsiasi altra Nazione ad economia sviluppata. Intendo far riferimento alla tempestività che una nuova normativa deve avere oggi per seguire ed adattarsi via via allo sconvolgimento finanziario intervenuto dopo il 15 settembre, dopo il fallimento della Lehman Brothers. Siamo ormai abituati a queste date: l'11 settembre, 15 settembre è un'altra data importante che non potremo dimenticare. Ma forse, più che di tempestività è bene parlare di giustapposizione delle leggi alla mutevole realtà economica e finanziaria che si va manifestando, ovvero l'economia reale nella attuale preoccupante congiuntura. Così, mentre è risultato di grande lungimiranza politica l'intervento triennale proposto dal ministro Tremonti e approvato dal Parlamento il mese di luglio scorso, oggi è assolutamente necessario il nuovo intervento, cioè il disegno di legge che prevede le nuove disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, vale a dire la legge finanziaria 2009. Certamente, la portata innovativa di questo disegno di legge può risultare riduttiva

La verità è che l'andamento della crisi finanziaria internazionale non ha ancora esaurito i suoi effetti negativi. E' difficile restituire fiducia ai risparmiatori (e in questo senso va considerato il decreto cosiddetto salva banche recentemente approvato) ed è ancora evidente la instabilità delle Borse valori, da quelle quelle asiatiche a quelle europee e nordamericane, che alternano tutte ottimismo improvviso e successive ricadute. Abbiamo visto ieri l'effetto positivo che l'annuncio del piano Obama per il settore automobilistico ha provocato ha provocato sulle Borse, da Wall Street all'Europa, al quale ha fatto seguito oggi un quadro generale ben diverso. Lo spettro della disoccupazione è ancora presente e si manifesta, anche in Italia, con cassa integrazione della FIAT (ma avviene anche alla Renault) che copre l'intero periodo delle festività ed oltre. Ecco Ecco perché il disegno di legge finanziaria al nostro esame assume un particolare valore: è un modo concreto di affrontare il bilancio nella congiuntura che stiamo sopportando. E' un modo concreto di stare con i piedi per terra, perché se in linea teorica siamo tutti consapevoli, maggioranza ed opposizione, moderati e riformisti, che le regole del libero mercato vanno sempre rispettate, è anche vero che se GM, Ford e Chrysler dovessero ottenere cospicui sostegni da parte del Congresso americano, sarebbe poi molto difficile negare in Italia lo stesso aiuto alla nostra unica fabbrica

Tenuto conto di regolazioni debitorie, delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo di ricorso al mercato finanziario sale inesorabilmente ed è fissato, se si tiene conto anche dell'indebitamento all'estero, in termini di competenza fino a 260.000 milioni per l'anno finanziario 2009. Va sottolineato il fatto che le maggiori disponibilità di finanza pubblica che si dovessero realizzare durante il prossimo anno rispetto al Documento di programmazione economico-finanziaria sono destinate alla riduzione della pressione fiscale per le famiglie, per i percettori di redditi medio-bassi, per i lavoratori dipendenti e per i pensionati. È questo un indirizzo prioritario del Governo, che esprime un'esigenza largamente avvertita in questo momento di disagio sociale. Certo, molto dipenderà dall'andamento della domanda interna e dalla crescita dei consumi. Intanto, per il 2010 e per il 2011, il saldo netto da finanziare, e quindi il ricorso al mercato finanziario, sarà rispettivamente di 245.000 e di 225.000 milioni di euro. Equità sociale, pressione fiscale, economia di mercato, finanza pubblica, livello dei consumi interni e, non ultimo, il previsto contenimento del PIL: sono queste le ragioni che portano la finanziaria 2009 ad assumere un valore fondamentale. Siamo di fronte a un punto di svolta: fronteggiare la crisi e predisporre le condizioni per la ripresa. Bisogna riprendere la ricerca per un'economia di mercato non contro l'uomo, ma per l'uomo, come i grandi sostenitori dell'economia libera e di mercato hanno sempre luminosamente sostenuto, da Hayek a von Mises, a Einaudi, a Erhard sino al al recente premio Nobel Paul Krugman. Nella difficile ricerca di un equilibrio tra facilitazioni tributarie e incentivi di tipo particolare, il disegno di legge interviene in termini settoriali e perfino localistici, con un criterio generale che è certamente ispirato alla ricerca di una piattaforma comune degli interessi individuali. Stiamo cercando un equilibrio economico-finanziario collettivo, ispirato alla ricerca del bene comune. Al riguardo, voglio sottolineare l'importanza di alcuni emendamenti del relatore, approvati all'unanimità dalla Commissione bilancio, in materia di scuola, deroga al patto di stabilità per interventi di sviluppo infrastrutturale e proroga del divieto per Regioni ed enti locali di stipulare contratti relativi agli strumenti anche un altro emendamento, che ha avuto lo scopo del tutto condiviso di tutelare importanti settori economici, come quello dell'ippica e più in generale del Comitato olimpico nazionale; esso mette però a rischio la capacità di alcune imprese di stare sul mercato, destinandogli l'intero aggravio fiscale, che dovrà essere sostenuto dal settore delle *new slot*. Mi auguro, comunque, come abbiamo detto in occasione dell'approvazione del precedente disegno di legge in materia, che il disegno di legge preannunciato dal sottosegretario Giorgetti, nel disciplinare tutta la materia dei giochi *on-line,* possa armonizzare il prelievo tributario su tutto il settore. Con la finanziaria 2009 si confermano le finalità già approvate a luglio e si realizza un intervento legislativo che è destinato ad avere effetto immediato nell'arco di tempo che corrisponde al bilancio dello Stato dell'anno che sta per iniziare. Mi avvio velocemente alla conclusione. Vorrei ricordare anche alcuni degli interventi previsti nel prossimo disegno di legge, quello cosiddetto anticrisi, perché credo che nessuno di questi provvedimenti possa essere considerato È evidentemente una serie di provvedimenti, quello di luglio, la finanziaria, il decreto salva banche, lo stesso federalismo fiscale e quello sul quale la Camera inizierà l'esame prossimamente, che hanno evidentemente evidentemente l'obiettivo di rimanere strettamente legati a questa situazione particolare. È allora importante sottolineare l'introduzione del pagamento dell'IVA al momento dell'incasso, così come è stato importante anche È importante sottolineare che è stato possibile attuare tutte queste rilevanti misure solo dopo aver concretizzato aver concretizzato interventi sulla solidità dei conti pubblici e delle banche. L'intendimento del Governo è quindi quello del rilancio dell'economia. In conclusione, desidero ringraziare per l'importante lavoro i relatori, i senatori Pichetto Fratin e Saia, il Presidente della 5a Commissione ed il sottosegretario Vegas. Credo che dobbiamo impegnarci nella ricerca di una più aggiornata cultura economica, economica, di una più elevata morale, di un sempre maggiore senso di responsabilità da parte sia della politica che del*management*. Se riusciremo a fare dei passi importanti in questa direzione

Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, confesso che è assai difficile misurarmi con questa finanziaria in quanto mi appare francamente assolutamente fuori centro rispetto alla situazione economica in atto, già assai pesante, e a quella che si prospetta nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, decisamente drammatica per le condizioni di milioni di donne e di uomini nel nostro Paese. Questa finanziaria non si misura, infatti, con il quadro economico in atto e in divenire; non fa i conti con i dati del Fondo monetario internazionale, che testimonia di una caduta pesante del PIL quest'anno e l'anno prossimo, nè tanto meno con le valutazioni dell'OCSE, che sono ancora più drammaticamente peggiorative; e non fa i conti, anzi si disinteressa, della situazione materiale di milioni di famiglie e di lavoratori. Il Presidente del Consiglio parla di ottimismo, incita ai consumi, invita a non spendere meno, in occasione del prossimo Natale, di quanto si sia speso l'anno scorso e con ciò esorcizza i dati i dati che ci fornisce il CENSIS, che testimoniano che il 44,7 per cento delle famiglie è - davvero - pessimista per l'immediato futuro, ne ha paura, non è in grado di valutare cosa succede, ma sa che qualcosa succederà di pesante e di grave; e che il 17,4 per cento dichiara di essere incerto e disorientato. Allo stesso modo, forse non sa, o preferisce non sapere, che 279.000 famiglie hanno difficoltà a pagare il mutuo e che

Stiamo parlando di redditi di persone in carne ed ossa, di 3.100.000 famiglie che hanno contratto debiti per l'acquisto di beni di consumo, cioè per arrivare alla fine del mese. Questa è la realtà, signori della maggioranza e del Governo, questa è la traduzione di quel «non si arriva a fine mese» così diffuso nel sentire comune degli italiani, che però pare non essere accettabile alle orecchie del Presidente del Consiglio o che, al più, lo porta ad immaginare che possa essere sufficiente intervenire con uno strumento di contrasto alla povertà quale quello della *social card*. Per quanto mi riguarda, assicuro che non ho alcun atteggiamento snobistico o superficiale rispetto a questo intervento di natura assistenziale, anche se avrei preferito avvenisse in maniera diversa. Contesto la forma, che considero vergognosa, della *social card* e mi piacerebbe che, invece, questo Paese potesse essere dotato di una legge di contrasto alla povertà che sappia sviluppare politiche sociali importanti, tese al reinserimento di chi si trova in condizioni di povertà assoluta. Il CENSIS ci parla del reddito delle famiglie, delle loro ansie, delle difficoltà, delle paure per la loro condizione materiale di oggi e di domani. Ma che dire della condizione del mondo del lavoro? Non meno di 10.000 imprese dell'industria, dell'artigianato e dei servizi sono coinvolte già oggi nella crisi. L'andamento della cassa integrazione guadagni, ordinaria, straordinaria e in deroga, e la gestione dell'edilizia, da gennaio a novembre, dimostrano la straordinarietà della crisi - insisto - già ora in atto. E se questi sono i dati del 2008, non so immaginare cosa capiterà nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Le ore di intervento di cassa integrazione sono state 280 milioni, con un incremento esponenziale negli ultimi 2-3 mesi: quindi, è qui il segno di quanto di quanto morda la crisi in queste settimane. Ricordo, solo a me stesso, che chi sta in cassa integrazione guadagna meno di 800 euro al mese. E si badi, stiamo parlando di lavoratrici e di lavoratori occupati a tempo indeterminato, ma poi - anzi, direi prima perché sono i più esposti e i più deboli - esistono le molte lavoratrici e lavoratori precari, in particolare quelli a contratto a tempo determinato, a *part time*, i collaboratori, i Co.co.co., i Co.co.pro., un vero e proprio esercito di persone che rischia il posto di lavoro. È con questo quadro che bisogna misurarsi e con questa necessità di fare un intervento pesante su due fronti, uno è quello della politica dei redditi e l'altro è quello degli ammortizzatori. Bisogna avere coraggio, bisogna immaginare di uscire da questa crisi in avanti, immettendo elementi di cambiamento, di tutele oggi, ma di cambiamento. Pertanto, bisogna avere il coraggio di giocare un punto di indebitamento del PIL sui redditi e bisogna immettere in questo Paese un sistema di ammortizzatori sociali universale,

E alla fine, signor Presidente, mi consenta di ricordare in quest'Aula che anche oggi, oltre ai 986 morti sul lavoro dall'inizio dell'anno, ci sono stati altri tre morti:

Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Sottosegretario, lo hanno ribadito anche gli altri colleghi: questa è una crisi tremenda, la crisi che sta toccando l'economia reale. Noi siamo in una fase di recessione e invece di varare una manovra che potesse attenuare gli effetti di questa crisi ne abbiamo varata una che che non aiuta a risolvere i veri problemi del Paese. Noi abbiamo una stretta creditizia, abbiamo imprese che sono strozzate dalle banche, abbiamo 3 milioni e 200.000 famiglie indebitate con mutui a tasso variabile, abbiamo tanti altri problemi e, mentre negli Stati Uniti Obama, in Francia Sarkozy, in Germania Angela Merkel, in Inghilterra Gordon Brown, in Spagna Zapatero, per attenuare gli effetti di una crisi economica che sta devastando gli assetti di quei Paesi impostano manovre per favorire politiche di sviluppo e nuova occupazione, voi, onorevoli rappresentanti del Governo e della maggioranza, imprigionati al moloc del decreto n. 112, dopo aver regalato tre miliardi di euro di ICI a chi non ne aveva bisogno ed altrettanti ai capitani coraggiosi, dopo avere accollato i debiti alla fiscalità generale mi riferisco ad Alitalia - avete messo in piedi una manovra che non tiene in alcun conto degli effetti gravissimi di questa crisi finanziaria che sta mangiando l'economia reale, falcidiando centinaia di migliaia di posti di lavoro. Non ci sono solo gli allarmi lanciati dalle organizzazioni sindacali che denunciano l'inadeguatezza delle misure del Governo a fronteggiare la crisi e la carenza degli ammortizzatori sociali. Basta dare un'occhiata in giro ai negozi vuoti ed al monitoraggio di alcuni istituti di ricerca per verificare il disagio sociale di vasti strati della popolazione, specie di quel ceto medio che non arriva neanche più alla seconda settimana del mese e deve indebitarsi per sopravvivere; quel ceto medio che nel 2002, lavorando in due in una famiglia, riusciva a vivere ed oggi, invece, ha dovuto tagliare tutto, anche i consumi necessari, anche i consumi alimentari. Non parlo dei consumi culturali: non si va più a teatro, non si va più al cinema.

Basta girare tra la gente, signor Sottosegretario, nei mercati, nei mezzi pubblici, come faccio io, come facciamo noi, per avere testimonianza diretta di una grave crisi economica, anche nel ricco Nord-Est e nei settori più produttivi, come la Brianza.

Si tratta del 31 dicembre. "Tiriamo avanti fino alla fine dell'anno - dicono alcuni imprenditori - poi decidiamo che cosa fare: mettiamo tutti in cassa integrazione o, magari, chiudiamo proprio la fabbrica e ci ritiriamo dagli affari. Molti di noi ormai hanno ordini in portafoglio per tre giorni, qualcuno addirittura non ne ha proprio, nemmeno per mezza giornata"». È probabile insomma che all'inizio del 2009 ci sarà un incubo,

Cina e India, arrivano più. Portafogli, ordini ormai vuoti, acquirenti che non pagano, concessionari e rappresentanti che dalla sera alla mattina scompaiono: insomma, un rituale che è ben conosciuto. poi quegli imprenditori che, anziché riempirsi di BOT e di utili, hanno puntato sulla crescita continua e hanno investito tutto quello che avevano nei capannoni e nelle macchine: adesso le macchine si stanno per fermare, dai capannoni non esce più niente e le banche sono davanti alla porta a richiedere loro il rientro degli affidamenti. Stanno per pagare cara la crisi anche i più svegli, quelli che avevano investito in Lehman Brothers e in Merill Lynch. Fino ad agosto giravano sulle loro Mercedes e raccontavano dei loro favolosi guadagni. Adesso rischiano di perdere anche la Mercedes. L'Eldorado sembra finito, sfumato e scomparso. E non si sa se tornerà ancora. E mentre in America Barack Obama, dopo aver vinto le elezioni, mette in cantiere una manovra economica espansiva per creare milioni di posti di lavoro, investe centinaia di miliardi di dollari nelle fonti energetiche alternative e nella difesa dell'ambiente, il vostro Governo litiga in Europa per rinviare alle calende greche gli adempimenti previsti per la tutela dell'ambiente e taglia perfino i finanziamenti già previsti per il risparmio energetico, addirittura con effetto retroattivo, penalizzando non solo le famiglie che avevano puntato su tali incentivi, sostituendo ad esempio la caldaia, cambiando gli infissi, scegliendo il solare termico o i pannelli fotovoltaici, o ristrutturando la propria abitazione per migliorare l'efficienza energetica,

basandosi sugli ecoincentivi che erano stati previsti nelle scorse finanziarie. Inoltre, mentre ritiene di combattere gli effetti della crisi, basando il rilancio dei consumi sulla carta di carità di 40 euro al mese (soldi benvenuti per tantissime famiglie, che però non servono a rilanciare i consumi), delibera ulteriori pasticci fiscali, come denunciato dalle Acli. infatti, penalizzati i nuclei con più figli, mentre la riduzione del 3 per cento dell'acconto IRES e IRAP per dare ossigeno alle imprese vale solo per un mese perché, a fine anno, le aziende dovranno restituire lo sconto. Insomma, onorevoli colleghi, più che una partita di giro, sembra una partita di raggiro, uno *spot* pubblicitario neppure ben riuscito. Per attenuare gli effetti di una manovra economica sbagliata e regressiva, noi dell'Italia dei Valori avevamo presentato una serie di emendamenti migliorativi: dalla riduzione dei costi della politica, con l'eliminazione della cumulabilità dell'indennità della carica di ministro con l'indennità parlamentare, alla riduzione dei rimborsi elettorali dei partiti politici; alla soppressione della legge mancia che mi risulta ancora presente nella manovra; dall'incremento dei fondi per le politiche della famiglia, delle politiche sociali dei fondi per alloggi e residenze per gli studenti universitari

Avevamo previsto anche un incremento del fondo per gli interventi straordinari di edilizia scolastica. Avevamo chiesto, signor Sottosegretario, una manovra coraggiosa: un pacchetto da 33 miliardi di euro - come stanno facendo tutti gli altri Paesi - non la piccola aspirina che non serve.

Per aiutare le famiglie, avevamo proposto un aumento del fondo per le non autosufficienze; una riduzione dell'imposta di registro sulla compravendita degli immobili (portandola dal 7 al 3 per cento e dal 3 all'1 per cento

cento. Avevamo proposto, quindi, di restituire potere d'acquisto a chi soffre, ai lavoratori e ai pensionati. Avevamo chiesto un aumento del 10 per cento delle detrazioni dei mutui prima casa. Signor rappresentante del Governo, signor relatore, lavorato insieme in Commissione bilancio e abbiamo combattuto per questi emendamenti. Infine, rispetto ad un Governo "liberista", avevamo anche chiesto di incrementare i finanziamenti falcidiati dell'Antitrust, ossia quell'Autorità che opera con meno di 300 dipendenti (mentre la Banca d'Italia ne ha 8.000) a garanzia della concorrenza e del mercato in settori delicati a tutela dei consumatori. A tal proposito, ricordiamo il provvedimento dell'Antitrust

così come ha rinviato alle calende greche la legge sulla *class action*, formidabile strumento a presidio delle buone regole su correttezza e trasparenza delle imprese, dimostra allergia alle regole, ritenendo che le logiche del *Far West* siano migliori per i cosiddetti *animal spirits*, gli spiriti animali, e per i mercatisti della domenica. Per queste ragioni, signor Presidente, non possiamo votare una finanziaria sbagliata che produrrà gravi danni all'economia, ai lavoratori, ai pensionati e a milioni di famiglie

*(PdL)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Sottosegretario, in questo periodo di forte crisi dei mercati finanziari si sente dire da tutte le parti politiche che occorre sostenere l'economia reale e, in particolar modo, quel tessuto produttivo che caratterizza il nostro sistema economico, costituito di piccole e medie imprese che, a loro volta, lo tengono in piedi. A queste affermazioni non sono seguite però, fino a questo momento, scelte di politica economica che realmente perseguano con coraggio la finalità di sostenere questo sistema imprenditoriale, favorendone la crescita e soprattutto mettendolo al centro dei programmi di intervento. In un contesto in cui la domanda interna diminuisce nel tempo

2007), in un contesto in cui le banche hanno aumentato il costo del credito, gli ordinativi si riducono ed è in crisi anche il mercato internazionale, le scelte di politica economica auspicabili dovrebbero andare decisamente verso il sostegno alle piccole e medie imprese per garantirne la stabilità, la competitività e la continuità nel tempo. Al contrario, le politiche economiche finanziarie adottate finora dal Governo non si dimostrano adeguate perché non investono sul sistema delle imprese. Innanzitutto, la legge finanziaria non prevede alle Tabelle A e B, relative ai fondi speciali, accantonamenti relativi al Ministero dello sviluppo economico pregiudicando così qualsiasi iniziativa per interventi in favore dell'economia e delle imprese nel corso del 2009. Analogamente, non sono previsti stanziamenti per il rifinanziamento di norme recanti interventi di sostegno all'economia, classificate tra le spese in conto capitale. Numerosi sono i tagli e le rimodulazioni per gli stanziamenti già esistenti di competenza del Ministero dello sviluppo economico Oltre a ciò, dobbiamo sottolineare la mancanza di interventi adeguati al sostegno della domanda per il rilancio dei consumi delle famiglie e per rispondere alle necessità d'investimento delle imprese, tanto che in tal modo si rischia di pregiudicare ancora di più la ripresa della crescita e la possibilità di contrastare la perdita del potere di acquisto dei redditi da lavoro e delle pensioni. Cosa dovrebbe fare il Governo per avviare un percorso che consenta alle piccole e medie imprese, ai piccoli e medi imprenditori, di uscire da questa congiuntura negativa con la certezza di non essere soli? Anziché insistere, come fa il Governo, verso una progressiva restrizione del funzionamento dei crediti di imposta - l'esempio eclatante sono gli investimenti sul risparmio energetico o sulla ricerca e lo sviluppo sarebbe necessario e auspicabile incentivarli, rendendoli automatici ed eliminando tetti ed autorizzazioni. Come penseremo di sostenere gli investimenti nel settore in un momento in cui già c'è contrazione delle spese per investimento? Fissando ulteriori tetti al credito di imposta o affossandolo con meccanismi burocratici? Sul versante del credito alle piccole e medie imprese il nostro partito ha sostenuto con forza, già dall'inizio della crisi finanziaria,

Camera, già da una prima lettura appare inadeguato perché prevede a favore dei Confidi risorse molto esigue, rendendo inefficace la misura. Una delle difficoltà più grandi per il sistema delle piccole e medie imprese nel nostro Paese è il grave ritardo con cui la pubblica amministrazionepaga i suoi debiti. Occorre un'azione veramente veramente coraggiosa per superare questa *impasse* anche attraverso la previsione di meccanismi di compensazione tra debiti e crediti coesistenti nei confronti della pubblica amministrazioni. Noi abbiamo già proposto, nel corso dell'esame di altri provvedimenti che sono passati al vaglio di questa Camera, proprio un meccanismo di compensazione tra crediti e debiti nei confronti della pubblica amministrazione, che è assolutamente sostenibile; peraltro, è stato recepito anche in un ordine del giorno il primo il primo sottoscrittore è la senatrice Leddi. Nulla, invece, si è fatto per favorire la ripatrimonializzazione delle imprese che, in un periodo in cui ci sarebbe l'esigenza di fornire maggiori garanzie patrimoniali agli istituti di credito, dovevano poter contare sulla rivalutazione dei cespiti immobiliari. Si tratta, però, di un provvedimento che il Governo non ha favorito. D'altra parte, insistere sulla necessità di favorire gli investimenti in nuove tecnologie, ricerca e sviluppo, energia pulita da fonti rinnovabili significa anche indurre una maggiore flessibilità al patto di stabilità interno, consentendo l'anticipo dei progetti di investimento pronti ad essere sborsati in poco tempo, a partire dai programmi cofinanziati dall'Unione europea. Cosa dire dell'imprenditoria femminile e giovanile che sono scomparse in questo momento dai pensieri del Governo comunque, non sono oggetto di adeguata attenzione quando, invece, costituiscono una delle chiavi dello sviluppo economico del nostro Paese? Vogliamo creare le adeguate opportunità per favorirne la crescita? Anche sul versante delle politiche energetiche il Governo non ha ancora il coraggio di fare scelte adeguate che tengano conto dell'attuale stato di asimmetria di trattamento in cui si trovano imprese e consumatori. Occorrerebbe in questo momento eliminare gli oneri impropri che gravano sul costo dell'energia ed estendere alle singole imprese i benefici previsti per le imprese energivore e quelli previsti per il risparmio e l'efficienza energetica per ridurre le differenze rispetto alle imprese comunitarie. Non si può sostenere che il calo recente dei costi dell'energia, che è indifferenziato in tutti i mercati, sia da solo sufficiente a facilitare la vita delle nostre piccole e medie imprese che si trovano a competere in un mercato globale ove ogni asimmetria con i competitori internazionali diviene svantaggio competitivo. Un'ultima breve considerazione - breve solo per il tempo a mia disposizione - è volta al comparto del turismo, che sembra essere al momento tra i più dimenticati dal Governo: quali investimenti sono stati fatti in questo settore? Si crede che realmente possa costituire un volano di sviluppo per la nostra economia? Non dobbiamo dimenticare che proprio nel turismo troviamo esperienze di impresa giovane ed innovativa che valorizzano il nostro Paese e lo fanno crescere a livello internazionale. Cosa sta facendo il Governo per questo settore? Sinora abbiamo sentito solo dichiarazioni di intenti.

e, per ripartire, io credo sia necessario intervenire in misura efficace, sia sul fronte dell'immediato (legge finanziaria 2009) che nel medio e lungo periodo. Occorrono cioè interventi atti a segnare la discontinuità e la ripresa reale del sistema economico-produttivo. A me pare, invece, che questo Governo abbia provveduto solamente ad intervenire con tagli, mortificando lo sviluppo e lasciando spazio ad una deriva recessiva in atto con il rischio di una stagnazione e, perché no, di un pericolo, alle porte, anche inflattivo.

Il Presidente del Consiglio, onorevole Berlusconi, afferma che ci sono 16 miliardi di euro che verranno stanziati per interventi infrastrutturali.

Una somma, illustri colleghi, molto consistente, che è composta per 391 milioni da una riduzione delle spese correnti e per 2,441 miliardi da una riduzione

*transhipment*, ed il capitolo 1351, che attiene al Fondo per il finanziamento dei servizi pubblici di viaggiatori e merci sulla media e lunga percorrenza, laddove veniva previsto e stanziato per lo scorso esercizio un importo di ben 104 milioni di euro.

La riduzione riguarda il programma relativo ai sistemi stradali, autostradali e intermodali. Viene soppresso il capitolo 7486, che ha per oggetto le spese per interventi di ammodernamento e di potenziamento della viabilità secondaria esistente nella Regione Sicilia e nella Regione Calabria non compresa nelle strade gestite da ANAS Spa. Come è noto, tale risorse sono state utilizzate - per chi non lo ricordasse, ma è già stato detto - a copertura degli oneri derivanti dal decreto-legge n. 93 del 2008 che riguarda l'esenzione ICI sulla prima casa: manovra che non ha tenuto conto di una corretta perequazione della capacità contributiva dei cittadini, finalizzata semmai ad una mera ed inutile immagine elettorale. Continuando nella politica dei tagli, perché questo voleva essere l'argomento principale del mio intervento, ritengo corretto segnalare al Parlamento interventi ulteriori in un settore molto delicato e importante, quali sono le

di mobilità e sicurezza derivanti dai programmati lavori di ammodernamento dell'autostrada A3 nel tratto Gioia Tauro-Reggio Calabria e per il miglioramento della qualità del servizio di trasporto e sicurezza nello Stretto di Messina. Un'attenzione a sé merita il taglio della missione 19, che attiene al disegno di legge finanziaria; mi riferisco alla casa, all'assetto urbanistico, alle politiche urbane e al territorio.

registra una riduzione di ben 223,1 milioni di euro rispetto al dato assestato nel 2008. Qual è la conclusione della mia amarissima riflessione? II Gruppo Italia dei Valori ritiene che anche questa sia l'ennesima occasione perduta, ma non è banale, è la finanziaria. Esprimiamo pertanto un parere fortemente negativo. Il quadro che ci appare non solo è poco rassicurante, ma va verso la conferma di un *gap* infrastrutturale che vedrà nel 2009 una complessiva riduzione degli investimenti del 25 per cento ed una prospettiva nel triennio che - a dir poco - è densa di nubi e di grigiore. Cari colleghi, se questa è la finanziaria del 2009, se questa è l'alba, il giorno che deve venire tarderà sicuramente a sorgere.

se questa è l'alba, io dico che - al contrario - il buongiorno si vede dal mattino, quindi, secondo me, oggi è un bel giorno.

oltre che ai colleghi di maggioranza, anche a voi, colleghi di opposizione, che avete dimostrato di proporre soluzioni costruttive, magari non condivisibili, comunque vi siete posti in molte occasioni in modo costruttivo. i miei complimenti e ringraziamenti per la qualità del lavoro svolto in Commissione. Come già sottolineato dal relatore, un primo elemento caratterizzante dell'importante disegno di legge in esame è l'essere conseguente e coerente al decreto-legge n. 112 estivo e questo costituisce un'innovazione positiva; particolarmente apprezzabile, infatti, risulta evidentemente l'avvenuta definizione in quella sede dei saldi. Un secondo aspetto positivo è dato dalla corretta e opportuna stabilizzazione a regime di alcuni benefici per certe categorie che strutturalmente vivono e agiscono in situazione di concreta difficoltà. Questo atteggiamento serio elimina evidentemente quella che io chiamo la spada di Damocle che ad ogni finanziaria gli interessati di cui sopra dovevano partire e sopportare.

relative alla frequenza di asili nido, dove più che l'importo, in realtà abbastanza esiguo, vale il principio dato dalla stabilizzazione di ciò che si ritiene buono e giusto. E ancora, ne abbiamo un esempio al comma 11 a proposito dell'accisa per il gas naturale per combustione per uso industriale, nonché al comma 12, riguardo al gasolio da riscaldamento per le zone montane ed il credito d'imposta sulle reti di teleriscaldamento alimentato da biomassa ed energia geotermica. Ma un terzo aspetto di grande positività di questo disegno di legge è dato evidentemente dal non assomigliare ai provvedimenti in cui la regola era accontentare i vari partiti, se non addirittura i singoli parlamentari. parlamentari. Ricorderete tutti, non pochi mesi fa, la necessità di trattare con il senatore Pallaro; qui «l'assalto alla diligenza», come da più parti è stato sottolineato, non c'è stato. Non lo avrebbe permesso il contesto di grave crisi; non lo avrebbe concesso la provata serietà di questo Governo. Lodevole e degno di essere sottolineato è l'atteggiamento di grande responsabilità di Governo e maggioranza per il nuovo modo di affrontare la legge finanziaria, capace di lasciare da parte tutte le norme localistiche e microsettoriali o regolamentari, decidendo di affrontare esclusivamente i grandi temi.

perché occorre inevitabilmente consentire il raggiungimento del pareggio di bilancio nei tempi pattuiti - lo ribadisco, nei tempi pattuiti - e non, come suggerito,

Lo faremo perché occorre dare credibilità all'estero su quello che dovrà diventare il nostro Paese; lo faremo perché, se non possono crescere le entrate, a causa della crisi e della voluta diminuzione dell'imposizione fiscale, allora non rimane che spendere meno. È naturale. Ma come spendere meno? Innanzitutto, occorre analizzare la spesa: un Paese serio e moderno oggi dovrebbe spendere quanto più possibile in spese in conto capitale. Possibilmente dovrebbe aumentare la parte destinata agli investimenti, capaci, oltre che di realizzare maggiori infrastrutture, di offrire posti di lavoro creati dall'economia reale e non - come dice il mio collega della Lega Nord Garavaglia - dall'economia di carta costituita dalla fabbrica degli stipendi, qual è la pubblica amministrazione

detto e sottolineato - non si può abbassare la spesa corrente, se non si vuole dar luogo ad una serie cospicua di licenziamenti.

questo Governo. Se dunque non si può licenziare a man bassa, bloccare il *turnover* nelle Regioni che presentano percentuali scandalose di assunzioni nella pubblica amministrazione, deve essere considerata una regola per il futuro. Negli ultimi dieci anni, le amministrazioni centrali hanno aumentato le loro assunzioni di 105.900 unità e le amministrazioni locali di 21.000. Il rapporto tra dipendenti pubblici e totali occupati diverge moltissimo se si paragonano le Regioni settentrionali a quelle meridionali: ad esempio, mentre in Lombardia tale rapporto misura il 12,8 per cento, in Calabria lo stesso rapporto è pari al 29

un aumento inutile di assunzioni spesso non produce un aumento di servizi, bensì un aumento di burocrazia, con una diminuzione evidente di competitività. il ministro Tremonti ci ricordava come l'Italia *ante* 1971 avesse un livello di debito pubblico entro il 35 per PIL; ci ricordava come ogni anno vi fosse un sostanziale pareggio della parte corrente, a volte con una creazione di risparmi, i quali consentivano, insieme al corretto ed equilibrato indebitamento, di realizzare gli investimenti necessari al Paese. Ogni azienda che si rispetti agisce così: questo è il modo naturale che ogni azienda sana ha di comportarsi, altrimenti semplicemente fallisce. Oggi paghiamo le scelte scellerate dei decenni successivi ai primi anni Settanta. Il problema è che non si può più rimandare la cura. Se non si può spendere in conto capitale prima di ridurre la spesa corrente, occorre evidentemente tenere in piede e agevolare la realtà imprenditoriale esistente e gli investimenti privati in attività imprenditoriali.

abbassare o, meglio, razionalizzare le imposte dirette alle imprese, man mano che i conti pubblici lo consentano, soprattutto alle piccole e medie imprese. In particolare - e si potrebbe farlo fin da subito - sarebbe importante sarebbe togliere un po' di burocrazia. Non si può non ricordare che le imprese italiane pagano ogni anno circa un punto di PIL percentuale in burocrazia: 15 miliardi almeno di euro buttati in burocrazia. per cento dei costi di questa burocrazia sono pagati nel Paese dalle piccole e medie imprese e il 76,3 per cento da aziende con meno di nove addetti. per non fare la figura di essere colui che parla bene ma poi non fa nulla, anticipo la presentazione di due miei ordini del giorno che vanno proprio in questa direzione e per i quali mi aspetto grande sensibilità da parte del Governo e del relatore. Anzi, il mio impegno, considerato che vengo proprio dal mondo imprenditoriale, sarà, ad ogni provvedimento che mi consente la non estraneità dell'oggetto, di portare alla luce alcune problematiche nei vari settori imprenditoriali, soprattutto di quella che chiamo burocrazia omicida, ossia quella che ammazza aziende ed economia. Ad ammazzare l'economia, specialmente quella delle piccole e medie imprese, a disincentivare un professionista a scommettere su se stesso quando all'inizio la decisione se scommettere o no è molto difficile, non c'è solo la burocrazia, non c'è solo la crisi che stiamo in questo momento soffrendo a livello globale, ma ci sono anche strumenti impositivi non giusti e non corretti. Mi riferisco al legiferare in violazione dell'articolo 3 dello Statuto del contribuente e agli studi di settore, così come sono concepiti oggi. Troppo spesso i precedenti Governi hanno violato l'articolo 3 dello Statuto del contribuente. Lo scorso Governo Prodi ha abusato di tale violazione. Questa è l'occasione buona per sensibilizzare maggioranza e Governo attuale a non legiferare mai retroattivamente in materia fiscale. L'impegno è a non derogare mai a questo pilastro di giustizia e correttezza per distinguersi in virtù ed equità nei confronti di chi le tasse le paga. Quanto agli studi di settore, nella legislatura precedente sono stati usati come una vera e propria *minimum tax*, almeno questo è ciò che io e molti altri miei colleghi in Commissione abbiamo rilevato. Oggi occorre tener conto della presenza di una crisi importante e quindi, coerentemente, le aspettative che il fisco ritiene di avere nei confronti dei risultati economici delle partite IVA interessate devono essere limitate. A questo vorrei aggiungere un ragionamento logico che riguarda le giovani partite IVA, i giovani professionisti, i giovani artigiani e imprenditori che verosimilmente per i primi tre anni di attività devono costruirsi quello che chiamiamo "avviamento". come possiamo equiparare un'aspettativa di risultato di una partita IVA consolidata, forte di un avviamento pluriennale importante, con quella di una partita IVA nuova e priva di avviamento? Sembra una domanda retorica, eppure le nostre norme non evidenziano Per questa ragione la Lega Nord chiede (e vuole sensibilizzare in questa direzione ancora una volta il Governo) di esentare dagli studi di settore e dagli indici di normalizzazione le giovani partite IVA nei loro primi tre anni di attività. Quale ulteriore considerazione, affermo che vorrei non si dicesse mai che questo Governo non intende combattere il sommerso e l'evasione fiscale sul territorio. Certamente è una delle missioni, anche se non deve essere confusa con la criminalizzazione fino a prova contraria di chi non sia un lavoratore subordinato e dipendente, errore questo già commesso in passato. Occorre comunque tener presente che secondo lo studio Quintavalle la pressione fiscale apparente nel nostro Paese è del 43,3 per

Quindi, l'invito, evidentemente, è di andare a controllare *in primis* soprattutto dove questo fenomeno è radicato e percentualmente più sviluppato. Ma il Sud per poter uscire dalla crisi fa dovrà curarsi con un cocktail farmacologico preciso: dovrà riuscire nella bonifica dalle mafie e dalla malavita, dovrà ridurre lo stipendificio creato nella pubblica amministrazione, abbassare quindi le spese correnti e destinare le risorse a quanta più possibile spesa in investimenti di conto capitale. Il Sud dovrà aiutare il concretizzarsi del federalismo fiscale, in esame parlamentare in queste settimane, perché solo con la realizzazione dei valori riconosciuti nel provvedimento di cui all'Atto come anche il resto del Paese, da una situazione di crisi senza precedenti. Anche per quest'ultimo motivo l'auspicio è che tutti insieme, maggioranza ma anche minoranza, attraverso un'opposizione costruttiva e non un irresponsabile eventuale ostruzionismo, si riesca a non far deragliare un treno che questo Governo ha collocato sulle giuste Su queste rotaie scorrono i principi di equità, di razionalizzazione della spesa, di rigore nei conti, di risoluzione dei problemi più annosi, di copertura dei buchi, ma non *gratis* per chi li ha creati, di diminuzione di burocrazia, di imposizione fiscale, soprattutto il merito dell'aver iniziato a porre le basi al blocco della spesa corrente ricorrendo al blocco del *turnover.* Infine, un riconoscimento al lavoro in Commissione bilancio: si è lasciato il necessario spazio alla discussione di ogni senatore; un provvedimento evidentemente poco modificabile ha subìto alcune puntuali migliorie prevedendo e risolvendo sul nascere una nuova questione legata alle scuole e agli prevedendo nuovi criteri legati al Patto di stabilità, come trasversalmente auspicato dalle forze politiche, prevedendo un'assegnazione di fondi ai Comuni di confine con le Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome (quest'ultimo emendamento fortemente voluto e sostenuto dalla Lega Nord). Per concludere un'ultima considerazione: come ricordato dal senatore Morando, quando prendiamo in mano il Paese non siamo molto fortunati: dopo l'11 settembre, questa volta dobbiamo affrontare una crisi storica, ma non voglio neanche pensare cosa sarebbe potuto accadere se ci fosse stato ancora l'ex Governo Prodi. l'opposizione propone una manovra espansiva, rinviando la data del pareggio di bilancio al 2012, forse al 2013; se ci fosse ancora Prodi, alla faccia della manovra espansiva, ci sarebbero Visco e Tommaso Padoa-Schioppaa comprimere l'economia con le loro bellissime tasse o ci sarebbero i vari Pallaro o Pecoraro Scanio, pronti a evidentemente a spendere tesoretti o quel che comunque c'è. Mi sa che noi siamo sfortunati, ma almeno il Paese una fortuna l'ha avuta. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Sottosegretario, stiamo discutendo e successivamente voteremo il disegno di legge finanziaria 2009, un testo snello e caratterizzato da alcuni elementi di forte novità, frutto di quelle scelte economiche avviate già a giugno con quella che è stata definita la "manovra d'estate" e che ha caratterizzato la politica economica del Governo definendo gli obiettivi principali, sia rispetto all'impegno assunto in sede europea, volto al raggiungimento del pareggio del bilancio entro il 2011, sia rispetto alla consapevolezza che un Governo responsabile aveva l'obbligo di interrompere quella tradizione nefasta della politica di bilancio italiana che ha portato il Paese ad avere il terzo debito pubblico del mondo. Per la prima volta, come fatto rilevare da alcuni colleghi, viene ora introdotto il principio della triennalità, proiettando le scelte su un orizzonte temporale più ampio, ma cosa ancor più importante è il ritorno ad una finanziaria che si riappropria del suo contenuto tipico, abbandonando quel carico eccessivo dì disposizioni e decisioni che ne deviavano la sua funzione originale. Una finanziaria che si perdeva in quel minestrone di provvedimenti discontinui, frammentari, microsettoriali, localistici, destinati non ad occuparsi dell'interesse generale del Paese, ma a soddisfare esclusivamente qualche interesse particolare, ad accontentare qualche territorio o l'appetito dei singoli o di qualche corrente. Colleghi, questa non è la finanziaria dei particolarismi, non bisogna mettere in atto nessun «assalto alla diligenza», occorre modificare quell'approccio con cui ogni autunno si affrontava la legge di bilancio. Oggi, è fondamentale blindare il bilancio dello Stato in un momento di grave crisi economica mondiale; è indispensabile continuare a dare iniezioni di fiducia al Paese e risposte concrete agli italiani, ma non è certamente facile per nessuno intervenire in uno scenario così caratterizzato. Il Governo ed il ministro Tremonti si trovano tra capo e collo il peso di una congiuntura economica che definire negativa appare forse troppo restrittivo. Occorre affrontare le emergenze ed attivare tutte le iniziative utili al rilancio del Paese, dalle grandi opere al varo di una strategia energetica nazionale, dal piano casa al contenimento del costo dei libri scolastici, dall'abolizione dei *ticket* sanitari alla *social card*, che voi avete superficialmente snobbato non pensando a quelle fasce deboli che purtroppo sono presenti nel nostro Paese. Certo, questo non basta, ne siamo consapevoli tutti, e saranno in molti che, prendendo coscienza degli aiuti all'economia che il Governo ha già messo in essere, non avranno esultato come alla vittoria dell'Italia ai Mondiali; ma certamente una piccola-grande soddisfazione, un piccolo sospiro di sollievo in molti lo hanno già tirato. Colleghi, essere intervenuti tempestivamente ha però evitato il tracollo. Mettere in essere quelle misure per il rilancio della competitività del nostro sistema economico, l'attenzione riposta nei confronti di coloro che rischiavano di rimanere troppo indietro, il rafforzamento delle finanze pubbliche hanno fortunatamente evitato il peggio. E qui non si vedono solo le capacità politiche di questo Governo, ma emerge la presenza di figure professionali altamente qualificate, di economisti di grande livello internazionale di cui

dal Governo Berlusconi è una politica di bilancio restrittiva e affermate che il Paese richiede invece misure di tipo espansivo, ma spero di cuore che non vi riferiate alle stesse misure messe in atto dal precedente Governo, quando è stato aumentato il prelievo contributivo sui lavoratori precari, quando è stato ridotto lo stanziamento per la cassa integrazione, quando è stato deciso di aumentare gli estimi catastali, sui quali si pagano le tasse sulla casa, quando, aumentando le imposte dirette e, di conseguenza, il peso delle aliquote marginali, veniva tassato quello che gli italiani a fatica guadagnavano con straordinari e premi di produzione, o quando sono state cancellate le grandi opere in grado di assicurare sviluppo e occupazione a centinaia di imprese e lavoratori. Colleghi, questo solo per rinfrescare un po' la vostra memoria, magari intorpidita dal freddo invernale di questi giorni. C'è una gran bella differenza tra l'aver dimenticato e il far finta di non ricordare. Come sosteneva infatti un noto giornalista e scrittore: voler dimenticare il passato è come voler dimenticare la legge di gravità; si può fare un salto, ma chi lo fa deve, quando ricade, essere più attento di chi ha fatto soltanto un passo. Ebbene, colleghi, il presidente Berlusconi e il ministro Tremonti in particolare, passo dopo passo, stanno continuando a percorrere a percorrere le due direttrici sulle quali è basata la manovra economica del Governo: il riordino dei conti pubblici e gli interventi per favorire lo sviluppo e rilanciare il Paese. Purtroppo, però, dovendo ridurre il deficit, ma non volendo in nessun modo mettere ulteriormente le mani in tasca ai cittadini e far pagare loro nuove tasse, esiste una sola soluzione: quella di operare un politica di serio contenimento della spesa pubblica. È un sacrificio richiesto a tutti i Ministri, ai loro Ministeri e a tutte quelle diramazioni delle strutture dello Stato che devono contenere privilegi e razionalizzare le spese per trasformare l'Italia dal Paese degli sprechi nel Paese dell'efficienza. Questo è il nostro obiettivo. Certo, colleghi, non basta contenere la spesa pubblica ed occuparsi delle emergenze per rilanciare l'economia: bisogna continuare a perseguire una scelta economica frutto di una visione generale, che porti ad un rilancio vero del Paese che gli consenta di consolidare la sua posizione nel sistema della grande economia mondiale. Per questo - e mi rivolgo anche ai colleghi dell'opposizione era necessario abbandonare l'uso speculativo che in questi anni si era soliti fare della finanziaria, la predisposizione di tutti quegli emendamenti per chiedere qualcosa per quel territorio, per quella Regione, per quella singola impresa. Oggi serve senso di responsabilità, serve una politica in grado di prendere per mano tutto il Paese, da Bolzano a Reggio Calabria per arrivare alla mia Sardegna. Un Paese che deve diventare sempre più solidale, agganciando i vagoni lenti al treno veloce dello sviluppo. Questo Governo e questa maggioranza sono sulla giusta strada.

dei disegni di legge finanziaria e di bilancio annuale e pluriennale dello Stato, come abbiamo già sentito in diversi interventi ed in particolare nelle relazioni iniziali,

uno tsunami - in campo finanziario, ha dato una guida stabile e un indirizzo al nostro Paese e ai nostri cittadini.

godendo di grande autonomia e di entrate finanziarie importanti, determinano una grossa disparità tra gli operatori

portare tutti i cittadini allo stesso livello per mezzo del federalismo fiscale, quindi con quell'autonomia e quella gestione dei redditi prodotti a livello territoriale, con un Governo vicino alla gente, secondo il principio della sussidiarietà. in questo momento di transizione è importante cercare di limitare il *gap* esistente e

lo sblocco ed una considerazione particolare almeno per quanto riguarda gli investimenti, sottraendoli dal calcolo complessivo. Anche questo è un segnale importante di attenzione del Governo e della maggioranza per quanto riguarda gli enti locali e la piena operatività che devono avere per intervenire in favore dei propri cittadini, pur ovviamente in un momento di restrizione delle capacità

quanto nostri testimoniin termini di cultura, di tradizione, di economia e di efficienza. Vanno considerati certamente con attenzione, ma devono essere razionalizzate le spese.

voglio ringraziare il sottosegretario Vegas per l'attenzione con la quale ha seguito tutto il dibattito anche in Commissione. Può testimoniare egli stesso che c'è stato finora un confronto serio e vero.

Vi sono due diverse impostazioni in campo: noi pensiamo che in un momento come questo bisognerebbe tentare di attuare il più possibile una politica espansiva,

a casa in cassa integrazione). Insomma, sul tema della cassa integrazione e degli ammortizzatori, vogliamo continuare ad andare in deroga di fronte a un problema che assume queste dimensioni?

ma di fronte a una crisi come questa sarebbe necessario che l'Europa nel suo insieme giocasse un ruolo a fianco degli Stati Uniti e si ponesse sul loro stesso piano per proporre un piano al quale

l'investimento nelle energie rinnovabili è una delle priorità assolute di quel Paese. Investire nelle energie rinnovabili in questo momento potrebbe rappresentare molto per il nostro Paese

e noi abbiamo un'IVA che ci penalizza dai 3 ai 5 punti rispetto agli altri Paesi nostri competitori. Possiamo continuare ad andare avanti così? Ridurre l'IVA in questo caso certamente costa, ma quanto dà di beneficio dal punto di vista della lotta del rilancio di un settore strategico come quello del turismo nel nostro Paese?

l'Italia perde dal 20 al 25 per cento di competitività del sistema Paese nella movimentazione delle merci. Non abbiamo una grande area logistica e i porti e i sistemi ferroviari nodali del Paese sono mal collegati dappertutto. La movimentazione delle merci per un Paese come l'Italia, che è strategico verso il Medio Oriente o verso l'Oriente, sarebbe una questione decisiva e fondamentale. Noi abbiamo un sistema che non funziona. Vogliamo dare priorità a questi investimenti che vanno ad incidere in maniera significativa e determinante su uno dei fattori di competitività sui quali l'Italia perde rispetto a tutto il resto d'Europa? Le nostre merci quando arrivano alla distribuzione perdono circa il 22 per cento rispetto agli altri Paesi. Paesi. Bisognerà allora decidere che, se si fa un piano di investimenti, ci si dà delle priorità e priorità serie, che si rispettano, e si chiede a tutti noi di fare un lavoro di questo tipo. Così si potrebbe sbloccare per gli enti locali l'infrastrutturazione di secondo livello.

vorrei rispondere subito al senatore Mercatali perché ha inserito nel dibattito, anche se alla fine di questa discussione, molti elementi interessantissimi dal punto di vista delle strategie economiche

aiuteranno questa maggioranza e questo Governo a trovare più facilmente con l'opposizione un filo comune e un interesse diffuso e ampio all'interno di quest'Aula parlamentare rispetto ai temi strategici strategici e nevralgici che lui ha affrontato questa sera e che interessano anche ciascuno di noi. Come non ricordare che solo un anno fa che solo un anno fa si lavorava in questi giorni a una finanziaria che tutto faceva tranne quello che ha appena detto il senatore Mercatali? Le scelte che, invece, il Governo sta operando in materia di finanza pubblica vanno giudicate complessivamente alla luce dei vincoli imposti dall'ordinamento, ma soprattutto dall'attuale congiuntura economico-finanziaria. Il Governo sta facendo quanto è possibile in un quadro economico nazionale e internazionale difficile la recessione in atto sta peggiorando. Lo testimonia il deterioramento delle prospettive di crescita dell'economia formulate nelle più recenti previsioni di autunno dei principali organismi internazionali che evidenziano come tutte le economie avanzate siano destinate a risentire, nel 2009, degli effetti della crisi finanziaria, mentre segnali di ripresa - che ci auguriamo - sono previsti solo a partire dal 2010. Tale contesto rende certamente opportuna la scelta del Governo, più volte dichiarata nel corso dell'esame del provvedimento in discussione, intanto di voler mettere in sicurezza i conti pubblici, stabilizzando e consolidando il quadro complessivo di finanza pubblica, e su questo innestare interventi di politica economico-sociale, mediante specifiche misure di settore. il decreto-legge n. 112 è stata definita la scelta del Governo di rivitalizzare la legge di bilancio in senso allocativo e di tipizzare la legge finanziaria, nel senso di lasciare ad essa il compito di regolare quantitativamente le grandezze di finanza pubblica. Sebbene non possa ritenersi concluso il dibattito sui documenti di bilancio - vanno ancora approfonditi alcuni aspetti, va fatto di più sul versante dei meccanismi e della qualità della spesa la decisione assunta fornisce una risposta decisa alla richiesta di razionalizzazione degli strumenti di bilancio e delle modalità di decisione parlamentare in voga fino alla scorsa sessione, proveniente - ahimè - da tutte le forze politiche. Appare quanto mai strumentale, quindi, la critica al Governo, reiterata nel corso della discussione in Commissione, di non prevedere, con lo strumento in esame, interventi volti al sostegno e allo sviluppo dell'economia necessari a fronteggiare l'attuale congiuntura, come ha appena detto il collega Mercatali. questo, un ritorno a provvedimenti *omnibus*, di cui noi non sentiamo certamente la mancanza. Vorrei ricordare che solo dopo l'entrata nell'euro è stato ampliato il contenuto della legge finanziaria stabilito dall'articolo 11 della prevedendo la possibilità di introdurre aumenti di spesa o riduzioni di entrata finalizzati al sostegno dell'economia ed allentando i divieti in materia tributaria previsti dalla riforma contabile del 1988. Credo sia assolutamente condivisibile la scelta del Governo di puntare sulla stabilità dei conti pubblici. La Nota di aggiornamento al DPEF aveva previsto un rialzo, seppure contenuto, delle previsioni sul deficit per il triennio, mantenendo fermo l'obiettivo del perseguimento sostanziale del pareggio entro il 2011, come dagli accordi intercorsi in sede europea. Inoltre, il quadro di finanza pubblica fissato con l'approvazione del ha previsto un livello di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche pari al 2 per cento nel 2009, all'1 per cento nel 2010, e allo 0,1 per cento nel 2011; un rapporto tra debito pubblico e PIL entro valori non superiori al 102,7 per cento per cento nel 2010 ed al 97,2 per cento nel 2011. È in questo contesto che si inseriscono gli interventi previsti dalla legge finanziaria, che conferma il saldo netto da finanziare, peraltro migliorandolo, dai collegati ancora in discussione e dal recente decreto-legge n. 185, attualmente in discussione alla Camera, che contiene interventi di economia reale volti a fronteggiare l'eccezionale situazione di crisi internazionale. In linea con le condizioni - tra cui la tempestività, la temporaneità ed il coordinamento degli incentivi a carico dei bilanci degli Stati membri - previste dalla Commissione europea per l'attuazione del recente piano di ripresa, messo a punto in sede comunitaria, tali interventi recano effetti migliorativi sui saldi di finanza pubblica, sia con riferimento al saldo netto da finanziare che in termini di indebitamento netto. A noi appare poi del tutto condivisibile la prudenza del Governo nel non abbandonarsi a facili sforamenti sul disavanzo, come avrebbero voluto in molti, anche sulla scorta del giudizio espresso dalla Commissione europea sul piano che abbiamo citato, in concomitanza dell'eccezionale congiuntura internazionale e della recessione in atto. Tutti sono d'accordo sul ritardo infrastrutturale del Paese, senatore Mercatali, ma è necessario porre estrema attenzione a questa materia, che va affrontata in maniera sistematica. Non siamo nella situazione, ad esempio, della Francia dove appare possibile sostenere un peggioramento al 4 per cento del rapporto deficit/PIL, conseguente alle spese per infrastrutture annunciate dal presidente Sarkozy. Così come nessuno può essere contrario ad interventi immediati in favore di categorie svantaggiate o in favore di fasce sociali deboli. Si discute invece sulle forme e sulla sostenibilità. Vorrei ricordare a qualche collega che durante la discussione in Commissione ha cercato di accreditare l'idea che tali interventi non sarebbero nelle corde, prima ancora che nell'agenda, del Governo, che sono passati solo pochi mesi dalla sciagurata scelta dell'allora maggioranza (la maggioranza di cui lei faceva parte, senatore Mercatali) di eliminare lo scalone Maroni, consentendo il pensionamento anticipato di poche migliaia di lavoratori che ha assorbito, però, un ammontare rilevante di risorse che avrebbero potuto essere più proficuamente impiegate, magari in situazioni di emergenza come quella attuale. La legge finanziaria appare quindi complessivamente equilibrata nelle misure che contiene. Tra l'altro, non mi sembra che la discussione in Commissione sia stata a senso unico e si sia fondata esclusivamente sul *continuum* Governo-maggioranza. Più volte il rappresentante del Governo ha evidenziato come il dibattito si sia svolto su binari ben diversi dal passato e sia stato caratterizzato da uno sforzo comune per fronteggiare l'attuale crisi. Nelle poche modifiche proposte dalla Commissione referente al testo approvato dalla Camera dei deputati appaiono significative, a mio modesto avviso, le misure relative alle scuole paritarie e al Patto di stabilità. Con riferimento alle prime, va ricordato che il ripristino pressoché totale delle risorse, circa 120 milioni di euro, in favore degli istituti in questione costituisce una garanzia per l'esercizio della libertà di scelta in materia di istruzione. Voglio rammentare che le scuole dell'infanzia, una rete che rappresenta in tutti i territori, laddove è organizzata, il principio di sussidiarietà con un anticipo di decenni prima ancora della sua formalizzazione nella Costituzione italiana che è avvenuta nel 2001, sopportano ed accolgono il 70 per cento dell'infanzia in età prescolare, consentendo allo Stato di risparmiare risorse enormi, giacché il costo annuo sostenuto per ciascun bambino nelle scuole paritarie nelle scuole paritarie è di 2.700 euro, che sono suddivisi tra contributi statali, regionali, comunali, donazioni e rette pagate dalle famiglie; nelle scuole statali, invece, il costo annuo per bambino è di 4.000 euro ed è sostenuto interamente dall'erario.

il reintegro dei fondi destinati alle scuole paritarie tra le scuole dell'infanzia, che rappresentano, in alcune realtà locali, l'unica forma di servizio pubblico.

di servizi pubblici adeguati; adeguati anche a favorire quella partecipazione femminile al mercato del lavoro che in tanti auspichiamo. Relativamente al Patto di stabilità interno, con il concorso dell'opposizione, alla quale diamo atto, ne è stato definito un alleggerimento, volto a favorire gli investimenti in infrastrutture degli enti territoriali, mediante la mancata applicazione delle sanzioni previste per quegli enti che investono appunto in infrastrutture autorizzate dal Ministero dell'economia. Tuttavia, sarebbe auspicabile un ulteriore approfondimento delle regole che sovrintendono il Patto, più volte da tanti di noi definito molto rigido e un po' stupido. In altri termini, sarebbe importante riconsiderare alcune fattispecie di poste contabili, per altro frequenti, e modalità di computazione che non consentono comunque ai nostri Comuni ed enti locali di rispettare gli obiettivi da conseguire. Allo stesso modo, e proprio in considerazione dell'attuale situazione finanziaria, appare necessaria, a mio avviso, una riflessione più compiuta sulla possibilità per Regioni ed enti locali di stipulare contratti relativi a strumenti finanziari derivati e di rinegoziare i contratti derivati a seguito della modifica della passività al quale il contratto stesso è collegato. Ho il sospetto che oggi, in questo clima, in questa situazione, riteniamo giusto - così come abbiamo condiviso e votato solo qualche mese fa - impedire la nuova stipula di contratti derivati da parte degli enti locali; allo stesso tempo, nell'attuale situazione,

in condizioni diverse, con le banche spesso straniere che hanno proposto ai nostri enti locali questo tipo di contratti definiti derivati, ma che potrebbero definirsi anche in qualche altro modo, poter ridefinire e ricontrattare questo strumento che rischia di diventare un cappio al collo ai nostri enti locali peggio del Patto di stabilità. È stato un lavoro intenso quello della Commissione bilancio, che ha lavorato su un testo innovativo, razionale, asciutto, ma non per questo meno denso di contenuti; un lavoro proficuo assegnato ai relatori Pichetto Fratin e Saia, che ringraziamo, affinché anche in Aula si concluda l'esito di questo *iter* parlamentare con la costruttività

della manifestazione di quelle che possono definirsi le esigenze categoriali, territoriali e settoriali, ma che sono importanti e rilevanti per

la domanda è come le misure anticicliche possano anche essere strutturali. Era la domanda che si poneva il relatore di minoranza, il senatore Rossi, quando chiedeva

e mi auguro, anche come relatore di maggioranza, che queste sperimentazioni non siano una pura misura anticiclica, ma che siano davvero propedeutiche a disegni molto più ampi.

non sia su questi termini che si possa porre il discorso. Credo quindi che nel confronto fra due tesi di cura per quanto riguarda l'immediato e di strutturazione degli strumenti giuridici di questo Paese si debba fare una prima valutazione. A di come intervenire nella cura, c'è una scelta di percorso? I colleghi si renderanno ben conto che un Paese che rappresenta l'1,5 o il 2 dell'economia mondiale ha poche armi per dettare gli indirizzi; forse potrebbe farlo l'Europa con la somma delle forze, unificando e indirizzando tutti nella stessa direzione

oceano. La suddetta valutazione mi porta a ribadire quanto sia corretta la posizione assunta dal Governo, che ha fatto una prima scelta, quella di porre in sicurezza

La teoria dei consumi, che il professor Rossi conosce bene e meglio di me, è figlia anche di prova statistica e non solo di teorie o o esercitazioni dottrinali, ci spiega come un flusso di denaro generalizzato non non raggiunga lo scopo di stimolare la domanda; questa è anche una replica parziale all'intervento del collega Mercatali quando citava la parte che riguarda l'IVA. Solo il 30-40 per cento degli eventuali maggiori flussi generalizzati di denaro si trasformerebbe in spesa e quindi sarebbe un vero stimolo alla domanda.

di quasi 400 miliardi di euro del nostro debito pubblico necessiti di una fermezza di bilancio e di garanzie che il mercato richiede, ma per l'interesse del Paese,

indebitato, con una rigidità della spesa pubblica senza uguali e una carenza infrastrutturale che mina la competitività, non è possibile fare azioni strutturali che in questo momento genererebbero duplicazioni. Credo, colleghi senatrici e senatori, che il dibattito abbia messo in luce queste due posizioni, ma anche la giustezza

perché proprio in un momento come questo, con imprevedibili cambiamenti a livello mondiale, l'aver fermi i confini e

legato alla riforma che, per il secondo anno di applicazione, riclassifica il bilancio per missioni e programmi. E' un sistema che va riconosciuto e che ci ha offerto la possibilità di rendere più agevole la lettura del bilancio, forse ancor di più quest'anno rispetto all'anno scorso, ritengo che comunque vi siano margini di miglioramento sia nella leggibilità che nella trasparenza dei dati, come avviene per gli indicatori di *performance* e in qualche caso anche di flessibilità, per poter offrire quindi maggiore accesso alla politica e ai suoi interventi.

non si può continuamente avere il torcicollo. Però è inevitabile che anche guardando oggi il quadro generale non si possa fare la fotografia di questa legge di bilancio senza capire da dove veniamo, la pressione fiscale degli ultimi anni, l'aumento di spesa ereditato dalle due precedenti finanziarie.

legata al ruolo di opposizione e di maggioranza o se effettivamente sia una miopia politica o peggio malafede. Mi rivolgo al relatore di minoranza che ha richiamato più volte la mancanza di coraggio da parte del Governo:

non solo di navigazione a vista ma attento al rigore ed a mantenere questa barra dritta. Al di là di tutto, comunque, è inoppugnabile che questa legge di bilancio migliora la finanza pubblica di fronte all'Europa e di fronte all'Italia. All'opposizione vorrei dire che i sostegni alle classi meno abbienti e alle aziende non sono finiti con questi due provvedimenti. Come abbiamo detto, il decreto n. 185 sta già dando risposte, ma ci sono

la senatrice Bonfrisco ha parlato di prudenza, il senatore Pichetto Fratin di realismo, il senatore Saia di responsabilità e la senatrice Germontani di tenere i piedi per terra. Si tratta, sostanzialmente,

nuovo. Nella legislatura del 1994 ci pensò il progressivo sfarinarsi - in una legislatura che non mancava di elementi di novità, lo riconosco - della maggioranza che ci pose rapidamente con i piedi per terra. Nella legislatura del 1996 andammo all'euro soprattutto per motivi di finanza pubblica e non per cambiare il volto del Paese, con il risultato che, una volta raggiunto l'euro, ci mettemmo con i piedi per terra con grande entusiasmo. Nella legislatura del 2001

sullo scoglio dell'articolo 18 e poi naturalmente «tenere i piedi per terra» fu giocoforza. Nella passata legislatura del 2006, per tenere i piedi per terra si perse l'occasione di un buon andamento delle entrate fiscali per restituire ai contribuenti quanto era loro dovuto, e temo che l'argomento lo stiamo riprendendo pari pari in questa occasione. Non so come dirvi, è divertente, se così posso dire, che la maggioranza non si renda conto che i suoi problemi oggi sono esattamente la conseguenza del fatto che abbiamo tenuto i piedi per terra. Se oggi dovete correre a fare la *social card* è perché tutti i Governi che vi hanno preceduto, per tenere i piedi per terra, non hanno costruito un sistema capace di tutelare le situazioni di maggiore difficoltà sociale ed economica. Se oggi siete costretti a inventarvi ogni giorno una deroga alla cassa integrazione, di formati sempre diversi ed a geometria variabile, è esattamente perché, per tenere i piedi per terra, tutti i Governi che vi hanno preceduto non sono stati in grado di fare la riforma degli ammortizzatori sociali di cui avevamo disperatamente bisogno. Quindi, l'argomento del tenere i piedi per terra è molto pericoloso; vi consiglierei veramente di stare molto attenti ad usarlo, perché potrebbe farvi rimettere sulla strada delle legislature precedenti. Per concludere, non so quanti piedi per terra avesse messo l'Italia del dopoguerra; non so quanti ne avessero gli italiani che sono andati a

alla fine di questa legislatura, saranno passati vent'anni dal 1994 ed io inizio ad avere la netta sensazione che, a forza di mettere i piedi per terra, abbiamo dimenticato come si alza la testa.